Sospendo la seduta, che riprenderà al termine della Conferenza dei Capigruppo, convocata alle ore 10. *(La seduta, sospesa

una nuova finestra"). La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il nuovo calendario dei lavori fino al 18 marzo. Questa mattina sarà discussa la relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni La seduta sarà quindi sospesa per riprendere alle ore 14,30 con la discussione, fino alla sua conclusione, del disegno di legge recante delega in materia di contratti pubblici. A tal fine la seduta non prevede orario di chiusura. Il termine di presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 11,30 di oggi. Il calendario della prossima settimana prevede la discussione dei seguenti argomenti: relazione sull'attività svolta dal Copasir dal 1° gennaio 2021 al 9 febbraio 2022 che, secondo i precedenti, si concluderà senza votazioni; dalla sede redigente, i disegni di legge sulla valorizzazione delle produzioni alimentari locali (approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) e sui prodotti alimentari della filiera corta (approvato dalla Camera dei deputati); il decreto-legge cosiddetto sostegni-*ter.* Il calendario prevede, se necessario, una seduta anche nella giornata di venerdì 18 marzo. Si informa, infine, che mercoledì 23 marzo, alle ore 15,30, il Presidente del Consiglio dei ministri renderà al Senato comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 24-25 marzo 2022.

sulla domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche del senatore Armando Siri nell'ambito di un procedimento penale.

parlamentari ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea di respingere la richiesta dell'autorità giudiziaria relativamente alle intercettazioni del 15 maggio 2018 - progressivo n. 2521 e progressivo n. per la incerta ed implausibile configurazione del requisito della necessità e, in relazione alle telefonate progressivo n. 2618 del 17 maggio 2018, progressivo n. 5760 del 27 luglio 2018, progressivo n. 5997 del 4 agosto 2018, progressivo n. 6043 del 6 agosto 2018, progressivo n. 6044 del 6 agosto 2018 e progressivo n. 6090 del 6 agosto 2018, di respingere la predetta richiesta non sussistendo il requisito della fortuità e occasionalità. Chiedo al relatore, senatore Malan, se intende intervenire.

ad essa per quanto riguarda i dettagli, che sono sicuramente di interesse nell'esame di questo documento, sintetizzo brevemente la questione. Si tratta della richiesta di

Il provvedimento del tribunale richiede per l'appunto l'utilizzazione di tutte quante, ma non ha richiesto l'autorizzazione (ritenendole palesemente inutilizzabili)

classificato queste conversazioni come un'intercettazione indiretta, ma nella consapevolezza che si trattava di intercettare le telefonate di un senatore, cosa che ovviamente è contraria all'articolo 68 della Costituzione.

La sentenza n. 188 del 2010 della Corte costituzionale specifica che stabilire la necessità

il requisito dell'assenza di intento persecutorio e quello della necessità dell'atto, motivata in termini di non implausibilità. Va detto che nello stesso documento del tribunale di Trapani si afferma di aver trasmesso tutte le risultanze emerse nell'ambito del procedimento in relazione alla vicenda relativa all'emendamento

una serie di richieste in ordine all'utilizzabilità di intercettazioni che aveva fatto il pubblico ministero, e la motiva proprio perché, da un certo momento in poi, già secondo il gup, il gup, benché siano intercettazioni indirette, è evidente che l'obiettivo dell'indagine sia il senatore Siri, quindi questo argomento è entrato nella motivazione del provvedimento al nostro esame. Vedo che il senatore Malan annuisce, perché giustamente ne ha dato conto anche nella sua relazione.

d'accordo con le conclusioni cui è giunto il relatore, ovvero che non si tratti più di intercettazioni casuali, perché è evidente che c'è ormai un'indagine mirata.

che sono comunque rilevanti, perché si sarebbe attivato nella sua veste di Sottosegretario. Ebbene, il relatore dice che al tempo di quelle due intercettazioni il senatore Siri non era Sottosegretario, quindi c'è un'implausibilità della motivazione. Questo è l'unico passaggio nel corpo di tutta la motivazione che è stato preso in maniera molto letterale, ma basterebbe dire

in quanto sono rilevanti perché relative a una condotta tenuta in qualità di senatore e Sottosegretario. locuzione la ribadisce più volte, in particolar modo a pagina 14, dove cita

voglio tenere lontanissimo dalla mia argomentazione il merito di un processo che non ci deve interessare assolutamente e non c'è nessuna tesi sull'accusa da questo punto di vista;

della motivazione si fa riferimento a una condotta come senatore e - come dicevo - nelle conclusioni si dice che le predette intercettazioni sono assolutamente rilevanti per la valutazione dei fatti, in quanto dalle stesse emergono i contatti tra l'imprenditore e il parlamentare, finalizzate alla presentazione degli emendamenti,

quando si esaminano le motivazioni, queste vanno esaminate ovviamente nel complesso e anche secondo la logica del provvedimento di cui ci stiamo occupando. È chiaro che nelle conclusioni - anzi, prima della

la motivazione - e non poteva essere diversamente - fa riferimento alle condotte contestate in entrambi i capi di imputazione, dove pacificamente una parte riguarda anche l'attività di senatore. La motivazione fa riferimento a un contesto, a una ricostruzione dei fatti, che naturalmente non spetta a noi in questo momento indagare o ricostruire. Quindi, per tutti questi motivi, non ritengo che possa essere utilizzato il criterio della implausibilità e della illogicità, per poi trasportarlo sulla necessità, con riferimento alle due intercettazioni di maggio. Aggiungo che questo è un criterio non estraneo alle nostre valutazioni e voi, colleghi, vedrete che si presenterà in altre occasioni che arriveranno in Aula; per esempio chi vi parla a questo criterio ha fatto ricorso, ma più

da accogliere la richiesta di inutilizzabilità di quelle sei e, invece, considerare utilizzabili quelle due. Quindi, anticipo che formulerò una richiesta di voto per parti separate.

Presidente, il procedimento penale a carico del senatore Siri, che è all'origine della richiesta di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni telefoniche, riguarda due capi di imputazione inerenti a fatti relativi a presunte fattispecie di corruzione. Il pubblico ministero, probatori, ha richiesto l'utilizzazione di tutte le intercettazioni acquisite dal cellulare di un indagato non parlamentare. Condivido pienamente la scelta del giudice dell'udienza preliminare di Roma di aver effettuato un primo vaglio sulla richiesta del pubblico ministero, riducendo la sua domanda di autorizzazione al Senato solo in relazione alle intercettazioni antecedenti alla iscrizione del senatore Siri nel registro degli indagati - iscrizione avvenuta il 25 settembre 2018 così ritenendo quelle successive come atti di investigazione diretta nei confronti del parlamentare, pertanto giustificabili solo in presenza di una autorizzazione preventiva. il giudice ha compiuto una corretta e apprezzabile distinzione dal punto di vista procedurale, nel senso che ha chiesto l'autorizzazione del Senato solo per l'utilizzazione delle conversazioni ritenute occasionali, cioè quelle avvenute quando non erano ancora emersi elementi concreti dai quali desumere che la persona intercettata potesse essere un interlocutore abituale del parlamentare. Nella seduta del 16 febbraio 2022, la Giunta ha deliberato a maggioranza di proporre all'Assemblea di respingere la richiesta dell'autorità giudiziaria: relativamente alle due intercettazioni del 15 maggio 2018, pur ritenute occasionali per l'incerta e implausibile configurazione del requisito della necessità; in relazione a quelle successive, dal maggio ad agosto 2018, per la mancanza del requisito della occasionalità. Con riferimento al caso di specie, *melius re perpensa*, ritengo che non solo le prime due telefonate del 15 maggio 2018 - peraltro brevissime e nello stesso giorno - ma anche quella di appena due giorni dopo (la telefonata del 17 maggio), sono tutte e tre da considerarsi certamente imprevedibili, occasionali e fortuite. Nel ristretto arco di due giorni, come avrebbero potuto rendersi conto gli inquirenti che l'interlocutore "Armando" fosse un parlamentare e, valutata nell'abitualità dei rapporti con l'imprenditore Arata, sospendere immediatamente le captazioni e richiedere l'autorizzazione al Senato? La Giunta, nella relazione approvata e oggi all'esame dell'Assemblea, pur ritenendo occasionali e quindi fortuite soltanto le prime due intercettazioni (quelle del 15 maggio 2018), ciononostante ne ha negato l'autorizzazione sotto il profilo della incerta e implausibile configurazione del requisito della necessità, in quanto intercettate anteriormente alla carica di Sottosegretario che il senatore Siri ha assunto in data 13 giugno 2018. Una asserita contraddittorietà della motivazione creerebbe - secondo la relazione approvata - un margine rilevante di incertezza rispetto al requisito della necessità del mezzo di prova, come delineato dalla Corte costituzionale. Per denegare l'autorizzazione, la relazione si avvale pretestuosamente di un riferimento contenuto nell'istanza dell'autorità giudiziaria di Roma: si tratta di un titolo dato all'informativa della DIA di Trapani, e non del tribunale - com'è erroneamente scritto nella relazione - con cui si trasmettono le intercettazioni alla direzione distrettuale antimafia di Palermo. In questa intestazione è scritto e cito testualmente: «Vicenda relativa all'emendamento proposto dall'imprenditore Paolo Arata e sostenuto dal senatore Siri nella sua veste di allora Sottosegretario del MIT». Vorrei che fosse chiaro che si parla di un'intestazione, di un titolo dato dalla polizia giudiziaria a un documento conclusivo delle intercettazioni, iniziate fin da quando il senatore Siri era senatore e completate quando era Sottosegretario. Tale intestazione non può assolutamente sostituire la valutazione dei fatti, che spetta solo e solamente al giudice. Si trascura in proposito che la necessità di cui parla la Corte costituzionale va valutata in relazione all'ipotesi accusatoria, secondo la quale è irrilevante che il sostegno ad un emendamento legislativo in cambio di utilità (si parla di 30.000 euro) sia dato nella qualità di senatore o di Sottosegretario, dato che entrambi tali *status* hanno la facoltà politica e fattuale di intervenire. Tant'è che nel capo di imputazione si contesta il fatto nella duplice qualità di pubblico ufficiale, senza alcuna distinzione tra la carica di senatore e quella di Sottosegretario. Inoltre, nella motivazione della richiesta di autorizzazione, il giudice dell'udienza preliminare di Roma così letteralmente si esprime: «Le predette intercettazioni sono assolutamente rilevanti per la valutazione dei fatti. Le stesse appaiono strettamente rappresentative del contesto spazio-temporale in cui avrebbe operato il senatore e sottosegretario Armando Siri, a seguito della consegna o promessa di denaro nelle modalità e finalità illecite prospettate dalla pubblica accusa». Da tale motivazione si trae la necessità del mezzo di prova e la congruità e la plausibilità della motivazione. Proprio la Corte costituzionale, nella sentenza 188 del 2010, rileva che la valutazione circa la sussistenza in concreto di tale necessità spetta indubbiamente all'autorità giudiziaria richiedente e detta autorità è tenuta, quindi, a determinare in modo specifico i connotati del provvedimento e a dare adeguato conto delle relative ragioni con motivazione non implausibile, così come è avvenuto ed è stato ampiamente fatto nel caso in esame. L'argomento sostenuto dalla relazione non è quindi assolutamente condivisibile, ma addirittura capzioso oltre che irragionevole e fondato su elementi di fatto inesistenti, ed espone - questa volta sì - il Senato alla possibilità che il giudice dell'udienza preliminare sollevi un conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale. Come ho avuto modo di sostenere recentemente, penso che la disciplina che regola queste prerogative dei parlamentari necessiti di una rivisitazione. Mi sto adoperando per depositare al più presto un disegno di modifica della legge di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, inserendo anche quanto esposto nei giorni scorsi in merito alle innovazioni tecnologiche da equiparare alla disciplina delle intercettazioni casuali. Ritengo che tale iniziativa, attraverso una più precisa procedura da adottare da parte dell'autorità giudiziaria, possa essere utile a garantire una maggiore tutela delle prerogative parlamentari e a definirne meglio i confini.

riguardo alla parte relativa alle due intercettazioni di maggio; quest'ultime verrebbero ritenute non utilizzabili sotto il profilo della implausibilità della motivazione e, quindi, della necessità.

nell'architettura istituzionale e costituzionale, cioè la difesa non semplicemente delle prerogative; ma, entrando nell'ambito delle prerogative e dell'applicazione della Costituzione, stiamo nella cultura costituzionale della separazione tra i poteri dello Stato. Poiché credo - come ho detto più volte che sia un argomento sensibile, che tra l'altro nell'evoluzione della società subisce compressioni e sollecitazioni, è un ruolo delicato e, quindi, esercitarlo correttamente, con equilibrio, stando esattamente in questa concezione, significa in definitiva difendere le prerogative dei parlamentari e non esporle a forme poi di delegittimazione che rischiano di travolgere l'impianto. Detto questo,

a verbale - come si dice in altre sedi - in modo che venga considerata a tutti gli effetti parte importante dei lavori con riferimento a questo provvedimento, che la nostra richiesta e la mia conseguente dichiarazione di voto intendono significare che la relazione è da intendersi motivata con riferimento a quanto risulterà approvato nella parte dispositiva.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, appare francamente difficile avallare la proposta conclusiva del senatore Malan, volta a respingere la richiesta dell'autorità giudiziaria relativamente alle intercettazioni del 15 maggio 2018 - progressivo n. 2521 e progressivo n. 2523 - per la incerta e implausibile configurazione del requisito della necessità,

e progressivo n. 6090 del 6 agosto 2018, di respingere la predetta richiesta non sussistendo il requisito della fortuità e occasionalità. È difficilmente argomentabile sotto il profilo della mancanza del requisito della necessità in quanto già preliminarmente il giudice per le indagini preliminari, nel caso di specie, ha proprio effettuato un vaglio sulla richiesta del pubblico ministero, riducendo l'ambito delle intercettazioni da sottoporre alla domanda di autorizzazione. Già a monte del nostro esame non è stata avallata la richiesta di utilizzo di numerose intercettazioni, in quanto il giudice per le indagini preliminari ha ravvisato la natura proprio indiretta di tali intercettazioni. Dopo una scrematura così ampia, la conclusione che sulle prime due intercettazioni manchi il presupposto della necessità onestamente mi sembra offensiva nei confronti della ragionevolezza di quest'Assemblea. L'argomentazione utilizzata dal relatore circa la non titolarità, a quella data, della carica di Sottosegretario appare incongrua, in quanto il senatore Siri aveva comunque la qualifica di parlamentare e, in virtù di tale *status*, aveva presentato emendamenti che - secondo l'accusa - erano correlati alla dazione di una utilità. Si contesta nella relazione conclusiva che le motivazioni sottese alla richiesta di autorizzazione all'utilizzo delle prime due intercettazioni siano scarne. Sembra quasi che un procedimento penale incentrato sui reati di corruzione e concorso in corruzione non sia una motivazione sufficiente per consentire l'autorizzazione delle prime due intercettazioni, che sicuramente si contraddistinguono per la natura casuale. Ricordiamo - e non per inciso - che, nell'ambito del procedimento penale in corso, si contesta al senatore Siri all'epoca sottosegretario di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - di aver proposto e concordato, con gli organi apicali dei Ministeri competenti per materia, l'inserimento di provvedimenti normativi di competenza governativa di rango regolamentare (quindi il decreto interministeriale in materia di incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile) e anche di iniziativa governativa di rango legislativo (la cosiddetta legge mille proroghe, la legge di stabilità e la cosiddetta legge di semplificazione); ovvero di aver proposto emendamenti contenenti disposizioni in materia di incentivi per il cosiddetto mini eolico, ricevendo la promessa e/o la dazione di 30.000 euro da parte del signor Paolo Franco Arata, amministratore dell'Etnea srl e *dominus* della Solcara srl, amministrata dal figlio Francesco Arata (società operative in quel settore), il quale - secondo l'autorità giudiziaria - da tali provvedimenti avrebbe tratto benefici di carattere economico. Si contesta altresì allo stesso Siri, sempre nella duplice qualità di senatore e di Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in concorso con altri coimputati, di essersi attivato per ottenere un provvedimento normativo *ad hoc* che finanziasse, anche in misura minima, con differimento dell'intera copertura finanziaria negli esercizi finanziari a venire, il progetto di completamento dell'aeroporto di Viterbo, di interesse della Leonardo spa, per future commesse. Il senatore Siri avrebbe inoltre esercitato pressioni sul comandante generale della Guardia costiera, per operare una sostituzione di un responsabile del procedimento per alcuni appalti in essere all'epoca dei fatti. In conclusione, nonostante le accuse e la rilevanza delle stesse, per il relatore non sussiste il requisito della necessità. Giuridicamente e politicamente non possiamo che manifestare la più profonda contrarietà alle conclusioni della Giunta delle elezioni la Giunta ha sostenuto il diniego all'autorizzazione, presupponendo il mutamento di direzione dell'atto di indagine che si ha nel momento in cui gli inquirenti, a partire dalla polizia giudiziaria che sta operativamente effettuando le intercettazioni su incarico dell'autorità giudiziaria, si rendono conto del coinvolgimento da parte di un parlamentare e della conseguente necessità di richiedere l'autorizzazione per proseguire le captazioni, che assumono in questo caso natura indiretta. La Giunta ha rinvenuto il cosiddetto *fumus mutationis* dopo le due telefonate del 15 maggio del 2018. Ora non si comprende perché l'intercettazione del 17 maggio 2018 non possa rientrare, considerata la vicinanza temporale con le prime due date, fra le intercettazioni casuali. Infine, per tutte le altre intercettazioni, anche se si può ipotizzare la sopravvenuta conoscenza da parte degli inquirenti della natura di parlamentare di uno degli interlocutori, la richiesta dell'autorità giudiziaria deve essere parimenti accolta, attesa attesa la gravità delle condotte contestate al senatore Siri, la cui conoscibilità non può essere ridotta entro lo schema delle guarentigie parlamentari. Per tutte queste considerazioni annuncio il voto contrario alla relazione del senatore Malan del MoVimento 5 Stelle. In caso di votazione per parti separate, andremo a diversificare il voto a seconda della formulazione delle stesse.

per avere contezza di quello che andiamo a votare. Rispetto alla relazione della Giunta, fino alla parola «necessità»,

Il disegno di legge, di iniziativa governativa, consta di un solo articolo e reca una delega al Governo per adottare entro sei mesi uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici. Le finalità perseguite dal disegno di legge, composto da un unico articolo, sono quelle di semplificare, razionalizzare e riordinare la disciplina in materia di contratti pubblici, nonché di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione di quelle già avviate. Il disegno di legge elenca i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi e, tra questi, si segnalano la necessità di evitare il *gold plating*; la previsione e la ridefinizione in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti e del personale in esse operante; la semplificazione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie di rilevanza europea; la semplificazione delle procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi, digitali, in innovazione e ricerca, anche ai fini del conseguimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; la riduzione e la certezza dei tempi relativi alle procedure di gara e di stipula dei contratti e all'esecuzione degli appalti; la revisione e la semplificazione delle procedure relative alla fase di approvazione dei progetti in materia di opere pubbliche; l'incentivo al ricorso a procedure flessibili per la stipula dei contratti pubblici complessi di lunga durata; la semplificazione dell'estensione delle forme di partenariato pubblico-privato, con particolare riguardo alla finanza di progetto; l'individuazione dei contratti pubblici esclusi dall'ambito di applicazione oggettiva delle direttive europee e la semplificazione della disciplina giuridica ad essi applicabile; il divieto di proroga dei contratti in concessione, facendo salvi i principi per l'affidamento *in house* e la realizzazione della disciplina sul controllo degli investimenti dei concessionari e sullo stato delle opere realizzate; la realizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento dei contratti da parte dei concessionari; la razionalizzazione della disciplina dei meccanismi sanzionatori e premiali, finalizzata a incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti pubblici da parte dell'aggiudicatario; l'estensione e il rafforzamento dei metodi di risoluzione delle controversie relative al rimedio giurisdizionale. È stabilito che i decreti legislativi così adottati abroghino espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino e comunque quelle connesse incompatibili e rechino opportune disposizioni di coordinamento in relazione a disposizioni non abrogate o non modificate. L'approfondito lavoro svolto dalla 8a Commissione sul provvedimento in esame, iniziato nello scorso autunno, ha incluso un articolato ciclo di audizioni dei principali attori del settore e ha condotto all'approvazione di 83 emendamenti, che complessivamente hanno apportato circa trenta modifiche al testo. Tale attività emendativa è stata ispirata a un metodo condiviso in Commissione nelle prime fasi della discussione, volto a contemperare le esigenze di definire più puntualmente i principi e i criteri direttivi della delega, con la volontà di non appesantire eccessivamente il testo. Nel corso dell'esame sono emersi, in particolare, alcuni temi che hanno registrato un'ampia convergenza dei Gruppi di maggioranza, spesso anche con l'opposizione, in un dialogo proficuo con il Governo. In primo luogo, si è condivisa la necessità di favorire la partecipazione di micro, piccole e medie imprese, inserendo un'indicazione in tal senso già nel primo criterio direttivo e introducendo poi un criterio direttivo specifico volto a prevedere la possibilità di procedere alla suddivisione degli appalti sulla base dei criteri qualitativi e quantitativi; nonché il divieto di accorpamento artificioso dei lotti, in coerenza con i principi dello *small business act*, anche al fine di valorizzare le imprese di prossimità. Un altro tema che, dato il particolare momento storico non poteva non essere oggetto di particolare attenzione è quello della revisione dei prezzi. La formulazione su cui alla fine è stato possibile convenire reca la previsione dell'obbligo, per le stazioni appaltanti, di inserire, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, stabilendo che gli eventuali oneri derivanti dal suddetto meccanismo di revisione dei prezzi siano a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa. Altro tema su cui si è registrata ampia convergenza è stato quello del divieto per le stazioni appaltanti, con riferimento ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, di utilizzare, ai fini della selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, il sorteggio o altro metodo casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari o specificatamente motivate. Scorrendo l'articolato normativo, tra le varie modifiche apportate si segnalano inoltre le seguenti: con riferimento al divieto di *gold plating*, si è specificato che rimane ferma l'inderogabilità delle misure a tutela del lavoro, della sicurezza, del contrasto al lavoro irregolare, della legalità e della trasparenza. In merito alla ridefinizione del regime della disciplina secondaria è stato inserito un riferimento alle diverse tipologie di contratti pubblici. In materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, è stato inserito un riferimento alla modalità di monitoraggio dell'accorpamento e della riorganizzazione delle stazioni appaltanti e la previsione di specifici percorsi di formazione, con particolare riferimento alle stazioni uniche appaltanti e alle centrali di committenza che operano a servizio di enti locali. È stata poi inserita una nuova lettera volta alla promozione, nel rispetto del diritto europeo, del ricorso, da parte delle stazioni appaltanti, a forniture, in quella parte di prodotti originari di Paesi terzi che compongono l'offerta, che non sia maggioritaria rispetto al valore totale dei prodotti. Nuovi principi direttivi rispetto al testo originario riguardano la razionalizzazione e la semplificazione delle cause di esclusione, al fine di rendere chiare e certe le regole di partecipazione; la previsione, in caso di affidamento degli incarichi di progettazione a personale interno alle amministrazioni aggiudicatrici, della sottoscrizione di apposite polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale, con oneri a carico delle medesime amministrazioni; la definizione della disciplina applicabile ai contratti pubblici nell'ambito dei servizi di ricerca e sviluppo. Per quanto concerne la qualifica degli operatori, è stato inserito un riferimento all'adeguatezza dell'attrezzatura tecnica e dell'organico. La Commissione ha poi introdotto un nuovo criterio di delega, volto alla ridefinizione della disciplina delle varianti in corso d'opera, nei limiti previsti dall'ordinamento europeo, in relazione alla possibilità di modifica dei contratti durante la fase di esecuzione. Un'altra novità rispetto al disegno di legge originario riguarda la revisione della disciplina relativa ai servizi sociali, alla ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché di quelle ad alta intensità di manodopera, prevedendo, come criterio utilizzabile ai fini dell'aggiudicazione, esclusivamente quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La Commissione ha inoltre ritenuto opportuno menzionare nel testo gli accordi quadro, le concessioni di servizi, la locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità. È stata poi prevista la revisione del sistema delle garanzie fideiussorie per la partecipazione ed esecuzione dei contratti pubblici, prevedendo, in relazione alle garanzie dell'esecuzione dei contratti, la possibilità di sostituire le stesse mediante l'effettuazione di una ritenuta di garanzia proporzionata all'importo del contratto, in occasione del pagamento di ciascun stato di avanzamento dei lavori. In materia di concessioni, si è previsto che siano disciplinate le concessioni in essere e non affidate con la forma della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica, secondo il diritto dell'Unione europea, con specifico riguardo alle situazioni nelle quali sussiste l'obbligo, secondo criteri di gradualità e proporzionalità, e tenendo conto delle dimensioni, dei caratteri del soggetto concessionario, dell'epoca di assegnazione della concessione, della sua durata, dell'oggetto e del suo valore economico, di affidare a terzi, mediante procedure di evidenza pubblica, parte dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle medesime concessioni, garantendo la stabilità del personale impiegato e la salvaguardia della professionalità. Infine, è stato introdotto un nuovo criterio di delega, dedicato specificatamente alla semplificazione delle procedure di pagamento, da parte delle stazioni appaltanti, del corrispettivo contrattuale, anche riducendo gli oneri amministrativi a carico delle imprese.

come - ad esempio - l'aver espunto dal testo originario del Governo il criterio del prezzo più basso, del massimo ribasso, nelle aggiudicazioni delle offerte basate solo sul criterio del prezzo.

un altro tema importante visto che recentemente le Camere hanno modificato l'articolo 9 della Costituzione, intervenendo proprio su tale questione e inserendo il tema della tutela ambientale

Dal punto di vista della digitalizzazione, siamo intervenuti facendo inserire un riferimento esplicito alla banca dati nazionale dei contratti pubblici e al fascicolo virtuale degli operatori economici: una grande semplificazione che si offre agli operatori, perché ovviamente tutto ciò che è inserito nel fascicolo virtuale non può essere più richiesto dall'amministrazione aggiudicataria, e questo sicuramente agevola il percorso. È l'attuazione di una cosa in verità iniziata molti anni fa, che stiamo arrivando finalmente a raggiungere questo obiettivo di grande semplificazione per le imprese.

limite poi abrogato perché non coerente con le direttive comunitarie. Fare in modo che le imprese siano imprese che fanno i lavori, che hanno uomini e mezzi, è assolutamente fondamentale per evitare di

Per quello che riguarda poi il divieto di sorteggio, ricordiamo che nei vari decreti semplificazione è stata aumentata

È importante considerare che chi scrive il codice sappia cos'è un cantiere o come si fa una gara, quindi questa interazione è utile ed importante per raggiungere l'obiettivo, ma anche e soprattutto per rispetto del Parlamento vi è il doppio passaggio parlamentare che prevede, una volta che il decreto legislativo è stato emanato e arriva in Commissione, che la Commissione possa fare osservazioni ma anche porre condizioni e, nel caso in cui il Governo non intenda recepirle, deve giustificarne il motivo e ritornare in Commissione parlamentare. Vi è stata, insomma, la volontà di rafforzare in maniera importante il potere parlamentare di interagire sul codice degli appalti.

al lavoro che abbiamo fatto in Commissione, forse sono entrati troppo nei particolari, per una legge delega come questa, e quindi potrebbero essere anche cassati nella loro esposizione. Al di là delle battute,

cercare e trovare soluzioni che andassero nella direzione di un'utilità per il Paese. Devo altresì ringraziare il vice ministro Bellanova

non so se abbiamo fatto, colleghi, fino in fondo e completamente il nostro dovere, perché il testo è migliorato, ma credo il testo è migliorato, ma credo davvero che si potesse fare di più. Troppe volte c'è questo vincolo, che ormai ci portiamo dietro, perlomeno in questa legislatura, per cui il Parlamento in fondo è giusto che intervenga, ma il meno possibile. Credo che questo non sia in linea con quella che deve essere la nostra attitudine ad intervenire sui testi normativi che vengono portati alla nostra attenzione. Semplificazione e operatività: dobbiamo velocizzare le procedure per gli appalti. Questo è il tema del testo normativo che affrontiamo ed è quello che ci aspettiamo dai decreti che verranno emanati; ma non sarà facile, lo dico chiaramente: non sarà facile perché serve più coraggio e spero che questo coraggio lo si trovi quando si scriveranno i testi. Con il Piano

avremo una capacità - e aggiungerei un dovere - di spesa e di investimento che sarà cinque-dieci volte la normalità, che già ci vede in affanno.

Dopodiché, c'è l'affidamento tramite gara dei lavori e anche questa - salvo contenziosi - normalmente dura uno, due, tre anni e dopo cinque-sei anni ci troviamo davanti a un'opera che può veder partire i propri lavori ma che allo stesso tempo rischia di non essere più attuale. attuale. Dobbiamo misurarci con questo quando diciamo, confermiamo e ripetiamo che bisogna essere più coraggiosi. Dobbiamo superare questa grande, troppa diffidenza che manteniamo nella collaborazione pubblico-privato. Sembra che scriviamo i testi, perché alcuni strumenti esistono, quasi come se non volessimo che venissero utilizzati.

ed è uno strumento previsto dal codice ma non utilizzato perché non vengono fatte quelle modifiche che lo renderebbero utilizzabile. Quando dico che questi strumenti vanno resi utilizzabili prima che sia troppo tardi. È mia convinzione che, nel giro di uno o due anni, rincorreremo i privati e il loro contributo perché si possa attuare il PNRR; ma rischierà di essere troppo tardi. Dobbiamo partire ora, dobbiamo farlo ora prima che sia troppo tardi. Sì, è vero - è nelle intenzioni e spero anche nel risultato del nostro lavoro - dobbiamo restituire alle disposizioni del codice semplicità e chiarezza di linguaggio. tale ambito però il rapporto Governo-Parlamento è sì corretto, però, come dicevo prima, rischia di vedere ancora troppa resistenza a una vera collaborazione che la cosa sia grave, soprattutto nell'ambito di una delega qual è questa. Se, infatti, il Parlamento deve dire meno possibile quando deve dare indicazioni per l'attuazione di una delega al Governo, credo che non sia sulla strada giusta.

È previsto dalla legge che il Governo possa utilizzare il Consiglio di Stato per emanare provvedimenti legislativi, ci mancherebbe; anzi, io credo che sia uno strumento non solo utile, ma molte volte è stato davvero prezioso per la nostra legislazione. Il fatto che il Consiglio di Stato scriverà i decreti attuativi - il che, ripeto, può essere una cosa positiva - sinceramente non ho capito perché l'abbiamo scritto nel testo. testo. Il Governo lo può fare automaticamente e autonomamente: perché lo abbiamo scritto nel testo? Credo sia stato sbagliato inserirlo nel testo, anche perché anche a me risulta - c'è stata una discussione - che non sia mai accaduto che si sia delegata al Consiglio di Stato una competenza così importante scrivendolo in un testo normativo. Lo si faceva di fatto, è bene che sia così. Abbiamo fortunatamente come come Paese un Consiglio di Stato e quindi dei consiglieri di Stato tecnici davvero all'altezza della situazione, che esprimono grandissime capacità legislative ed è bene assicurarci che esse possano servire all'attuazione del nostro lavoro del nostro lavoro e quindi della normazione. Ripeto però che il fatto che si sia volutamente andati avanti confermando la presenza nel testo non ci piace. Non credo che ciò sia stato adeguato; l'abbiamo assunta come una richiesta chiaramente accettabile, ma non ci piace. Riteniamo che non vada nella direzione giusta anche perché comunque, quale che sia la lettura, è di difficile comprensione in un certo senso e non ci lascia tranquilli. Qual è infatti la lettura? Il Governo voleva assicurare il Parlamento che non avrebbe scritto i testi delegati?

legge; non mi sarei mai permesso infatti di presentare un emendamento che vincolasse il Governo a dover assolutamente e obbligatoriamente dare al Consiglio di Stato questa competenza che,

È fondamentale comunque raggiungere l'obiettivo e in questo la Commissione e il Governo hanno lavorato bene per arrivare nella direzione giusta e unica di costruire un provvedimento che possa dare le risposte che i cittadini, le imprese e il Paese ci chiedono. Confidiamo anche che nei prossimi sei mesi, nei quali verranno approvati i testi, si mantenga un rapporto costruttivo e collaborativo con il Parlamento, perché è nell'interesse di tutti e soprattutto nell'interesse del Paese. Certamente noi faremo la nostra parte.

esame delega il Governo, come hanno avuto modo di esporre anche in maniera molto ampia i relatori, ad adottare entro sei mesi

e della regolazione della spesa pubblica, ove pubblico e privato si trovano ad interferire contraendo delle obbligazioni, ognuno per le rispettive competenze e ruoli, per creare sviluppo, costruire infrastrutture, assicurare manutenzioni, servizi e forniture. Fino a un paio di decenni

limitato a elencare le principali norme che nei decenni più recenti hanno cercato di riformare e semplificare il sistema dei contratti pubblici istituito nuove regole di formulazione e gestione di detti contratti, delle procedure e del sistema stesso di qualificazione delle imprese, con cambiamenti anche radicali. Siamo passati dall'Albo nazionale dei costruttori, ai provveditorati e alle società organismi di attestazione Parafrasando il codice civile, direi che il contratto pubblico è un atto con il quale una parte (un privato, quasi sempre) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o un servizio verso un corrispettivo in denaro (e ciò, in questo caso, per un ente pubblico). È, in senso lato, una prestazione di lavoro autonomo, un'obbligazione a mezzo di impresa. Il contenuto della prestazione è dunque il compimento di un'opera o un servizio per la produzione di un risultato. Per opera intendiamo il risultato di un'attività di elaborazione e trasformazione di materia tale da costruire un nuovo bene, mentre per servizio una produzione di una utilità (quindi il risultato di un lavoro), senza elaborazione e trasformazione di materie. Più semplici sono le forniture, con una semplice cessione di materiali. Essendo il committente un ente pubblico, occorre però mettere in atto dei metodi che garantiscano *in primis* la trasparenza delle procedure e la concorrenza. L'obiettivo della riforma è principalmente quello di ridurre le norme e razionalizzare il settore dei contratti pubblici, armonizzando la disciplina interna con gli indirizzi comunitari. Ci sono diverse tappe già segnate: dalla revisione del codice dei contratti, al decreto attuativo conseguente, all'entrata in vigore di tutte le leggi, regolamenti e provvedimenti attuati per la revisione del sistema dei contratti pubblici, fino al pieno funzionamento del sistema nazionale dell'*e-procurement*. Stiamo parlando di una riforma organica che garantisca il confronto competitivo e lo snellimento delle procedure, *conditio sine qua non* per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Occorrono criteri chiari e inconfutabili per l'aggiudicazione delle commesse. Oggi accade sovente che i tempi relativi alle procedure di gara siano spesso allungati in maniera considerevole a seguito di ricorsi che nascono proprio da criteri riportati nei bandi e nei disciplinari di gara spesso troppo articolati ed esclusivi, piuttosto che inclusivi, pertanto si prestano facilmente a essere oggetto di contenzioso, quindi a essere contestati. Oggi l'informatizzazione e la digitalizzazione possono costituire una base solida sulla quale il sistema dei contratti pubblici può essere riformato nel migliore dei modi: un nuovo, più snello e meno oneroso sistema di qualificazione e procedure di aggiudicazione chiare e finanche veloci possono caratterizzare questo nuovo corso storico che ci apprestiamo a intraprendere, pandemia e malaugurati conflitti alle porte d'Europa permettendo. Norme semplici e regolamenti chiari sono alla base di ogni lavoro produttivo (che si tratti di un codice, una circolare, un bando o un disciplinare) e direi anche indispensabili per prevenire ricorsi e contenziosi. E qui occorre insistere anche sulle procedure concernenti l'approvazione dei progetti attraverso lo snellimento di ogni *iter* che rende cantierabile un progetto: impresa ancora oggi - mi duole dirlo - titanica per alcune tipologie di opere e in alcuni contesti, dove organi stessi dello Stato (centrali e periferici) sovente si contendono pareri e nulla osta. Una buona norma in questo settore è utile a ridurre la spesa improduttiva a carico dello Stato a ridurre il costo del lavoro, se si tagliano o si riducono dei costi che gravano sulle imprese senza un palese beneficio. Il semplice ritardo in un qualunque programma di investimento è già un costo costo per l'investitore e per la collettività tutta che beneficia di quel servizio o di quell'opera: stando alla storia più recente devo dire che la vedo dura, soprattutto a certe latitudini, dove occorrerebbe forse creare delle *task force* dedicate. Se scendiamo nello specifico, a titolo esemplificativo penso all'incentivazione delle procedure di *project financing,* al potenziamento di meccanismi di rafforzamento delle procedure di risoluzione delle controversie alternative alle cause civili, quindi al ricorso ai tribunali, ma soprattutto alla creazione di albi e di sistemi di qualificazione e criteri di selezione (bandi, disciplinari, procedure) in cui ci si possa avvalere dei nuovi strumenti che oggi le tecnologie informatiche ci offrono. Potrebbe essere il momento giusto ed un metodo ben un metodo ben studiato e concepito potrebbe essere lo strumento adatto per un'autentica e più dinamica modernizzazione di questo Paese e di tutte le sue strutture decisionali ed operative.

di rendere possibile ciò che soltanto qualche mese prima sembrava una mera utopia sul fronte delle politiche comunitarie. Con il Next Generation EU la Commissione europea diceva sostanzialmente addio ad anni ed anni di rigido rigorismo e a quell'ossessione quasi cronica sulle regolette contabili. La pandemia, scatenatasi all'inizio di quell'anno, ha costretto i vertici del nostro continente a invertire il paradigma economico, immettendo di fatto benzina nel serbatoio delle politiche espansive e favorendo un nuovo, massiccio piano di investimenti, al fine di consentire alle economie del vecchio continente di reggere l'urto spaventoso della crisi arrivata con il propagarsi del coronavirus. Da quella famosa notte estiva, come è ben noto a tutti, l'Italia è stato il Paese che è riuscito a portare a casa la fetta di torta più grande e da lì è partito il percorso che ci ha condotto al Piano nazionale di ripresa e resilienza, il classico treno che forse davvero passa una volta nella vita, destinato a diventare di fatto uno spartiacque nella storia politica, economica e sociale del nostro Paese. Nel fornirci, quindi, questa irripetibile occasione e opportunità, l'Europa è stata però perentoria nel fissare inequivocabili paletti lungo questo cammino e ha chiesto a chiarissime lettere all'Italia di abbandonare la sua atavica inconcludenza sul fronte delle riforme strutturali, che per decenni sono state sbandierate e spesso strillate nelle campagne elettorali, ma che poi sono rimaste lettera morta e spesso magari incagliate in beghe partitiche e politiche. Sul fronte della regolamentazione dei contratti pubblici eravamo già consapevoli dal primo giorno di questa legislatura che l'impianto del codice degli appalti uscito dalla riforma 2016 era sicuramente fallace, ma anche superato. Come MoVimento 5 Stelle, un lavoro profondo di rivisitazione lo abbiamo realizzato già prima del Covid-19, in particolar modo durante il primo Governo Conte con lo sblocca-cantieri e poi con il decreto-legge semplificazioni nel secondo Governo Conte. Due provvedimenti che, di fatto, hanno rimesso in moto la macchina dei cantieri delle grandi opere pubbliche nel Paese, completamente ingolfata di fronte all'insostenibile ginepraio burocratico creatosi negli anni. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha reso, però, necessario un ulteriore intervento, al fine di semplificare ancora di più i meccanismi normativi delle gare d'appalto, per consentire

Voglio essere sincera: da parte di tutte le forze di maggioranza e non solo, qui in Senato, a conferma del fatto che comunque la Commissione, quando lavora, lavora bene, c'è stata la massima disponibilità verso un approccio costruttivo su questo tema. L'ottima quadra trovata sul metodo si è poi riflessa anche sul merito, visto che abbiamo comunque portato a casa risultati considerevoli sul fronte della semplificazione, della trasparenza e della tutela ambientale.

È vero che tale coinvolgimento è sancito per legge da tempi remoti, grazie a un regio decreto del 1924. Un conto, però, è dare la possibilità al Governo di chiamare in causa il Consiglio di Stato, un altro è che ciò avvenga sostanzialmente di *default*, con un pericolo, che dovrebbe stare a cuore a tutto il Parlamento, ovvero quello della deresponsabilizzazione del Governo su una questione così decisiva. Noi riteniamo che, su una materia nevralgica come quella dei contratti pubblici, i ruoli di Parlamento e Governo debbano rimanere centrali e baricentrici. Su questo specifico punto dei risultati comunque li abbiamo portati a casa. D'ora in poi, qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari, sarà chiamato nuovamente a trasmettere i testi alle Camere con tutte le osservazioni del caso, per un ulteriore passaggio. Sempre in merito alla stesura da parte del Consiglio di Stato dei decreti attuativi, ci sarà l'obbligo di avvalersi di magistrati del TAR, esperti esterni, avvocati e rappresentanti dell'Avvocatura generale dello Stato, rigorosamente a titolo gratuito. Come sempre, si è lavorato per giungere a un compromesso sensato e non possiamo che ritenerci soddisfatti, perché tutte le forze politiche avrebbero ovviamente voluto qualcosa in più. Si è lavorato col buon senso in questa Commissione in Senato e ora avremo delle procedure molto più a misura di impresa, oltretutto senza ricorrere a quei criteri, molto pericolosi, del prezzo più basso e del massimo ribasso. Ci riempie sicuramente d'orgoglio l'obbligatorietà dei criteri ambientali minimi. Siamo pur sempre la forza politica che per anni si è battuta per inserire la tutela dell'ambiente nella nostra Costituzione, battaglia definitivamente vinta soltanto poche settimane or sono. Qui e ora ci preme far passare un paradigma, anche in vista del futuro, al di là dei doverosi rilievi costituzionali: Parlamento e Governo non vanno deresponsabilizzati o aggirati su una materia come questa, come su tante altre. *(Applausi)*.

Prima di entrare nel merito del provvedimento vorrei rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i componenti dell'8a Commissione che, con spirito costruttivo e con franco confronto, hanno affrontato il complesso tema della delega al Governo in materia di contratti pubblici. Soprattutto rivolgo un grazie speciale ai due relatori, la senatrice Pergreffi e il senatore Cioffi, che, ancor prima di essere rappresentanti eletti dal popolo sovrano, sono soprattutto espressione dell'architettura e dell'ingegneria civile, quindi sono dotati di grande competenza e professionalità. Il nostro contributo per semplificare la disciplina che regola i contratti pubblici ha l'obiettivo di garantire chiarezza e sostegno alle nostre attività produttive. Ho il grande onore di essere firmatario, insieme ai colleghi della Lega e di tutta la Commissione, di emendamenti che tutelano il *made in Italy* nelle forniture pubbliche, garantendo una quota maggioritaria di prodotti italiani rispetto a quelli di altri Paesi *extra* UE. Infatti, l'opportunità di rilancio offerta dai fondi europei e la situazione di crisi attuale delle nostre imprese avevano reso urgente un intervento, per limitare l'afflusso nei mercati europei di prodotti di provenienza extracomunitaria a basso costo e quindi di materiale scadente. Abbiamo chiarito e reso più comprensibili agli imprenditori le regole che configurano l'illecito professionale e i motivi che potrebbero escludere le aziende dai bandi. Con la particolare sensibilità che ci caratterizza come Lega sui territori, abbiamo ottenuto la possibilità di suddividere o accorpare gli appalti in lotti. Questo gioverà, sia sotto il profilo di una maggiore garanzia di accesso al mercato da parte delle piccole imprese sia sotto l'aspetto della tutela delle aziende operanti in un determinato territorio, valorizzando così quelle di prossimità. Anche per un altro emendamento c'è un successo, ossia per il vincolo obbligatorio per la revisione dei prezzi in situazioni particolari. Questo è un grande risultato per parametrare i costi al reale andamento del mercato. Questo rappresenta un sostegno importante per le imprese del territorio, che saranno così nella condizione di fronteggiare situazioni eccezionali e imprevedibili, come quelle che stiamo purtroppo vivendo da mesi. La revisione dei prezzi, infatti, durante l'esecuzione del contratto si rivela necessaria per mantenere reciproco l'equilibrio tra il contraente e l'esecutore e così dà la possibilità alle imprese di fare offerte congrue, salvaguardando il principio di sana e leale concorrenza. È passata, inoltre, nel corso dell'esame, una nuova disciplina del ricorso al sorteggio, che, grazie alla Lega, dovrà essere fortemente limitata e regolata, in quanto si tratta di un meccanismo che svilisce la qualificazione acquisita dalle imprese. Inoltre, siamo anche fieri di un emendamento approvato, che prevede siano a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi professionali a favore del personale impiegato dalle stazioni appaltanti, cosa che non era scontata. Così, i loro costi saranno a carico delle stazioni appaltanti medesime. Sono stati infine accolti anche due ordini del giorno della Lega e altri tre importanti della Commissione che, come Gruppo Lega, abbiamo sottoscritto. Essi prevedono, da parte del Governo, l'impegno a prevedere una revisione dei tariffari delle società organismo di attestazione, le cosiddette SOA, a valorizzare l'esperienza del direttore tecnico dei lavori, a disciplinare il tema dell'equo compenso per i professionisti impegnati nell'ambito dei contratti pubblici, a realizzare tempestivamente una piattaforma digitale italiana delle costruzioni e a provvedere alla semplificazione delle verifiche antimafia. Mi unisco alle parole pronunciate dall'amico, senatore Paroli, poc'anzi, perché è chiaro che il Parlamento, nonostante il lavoro che è stato fatto in Commissione e nonostante si siano ottenuti risultati concreti, deve ritornare a essere una parte attiva della legislazione e non deve derogare ad altri organi il compito per cui siamo stati eletti. Tuttavia, Tuttavia, posso affermare che siamo orgogliosi di aver portato a casa questi risultati, che sono concreti, frutto di trattative con la maggioranza e con il Governo. E sono risultati che la Lega non avrebbe potuto ottenere stando all'opposizione. *(Applausi)*.

la necessità di varare delle politiche efficaci di ripresa economica oggi ci porta a discutere di appalti pubblici, che da sempre costituiscono una leva fondamentale di politica economica e sociale. Proprio nella fase dell'emergenza Covid, il tema ha assunto una funzione essenziale essenziale e rinnovata di contrasto alla crisi, con la possibilità di immissione di liquidità immediata nel sistema produttivo. La ripresa e la resilienza quindi non possono non prendere in considerazione le problematiche mai risolte dalla normativa sugli appalti. È importante che, proprio nel contesto del PNRR, si sia deciso di intervenire per regolamentare la materia dei contratti pubblici con misure urgenti - conosciamo già i decreti approvati - e misure a regime. Proprio tra le misure a regime rientra la revisione dell'attuale disciplina del codice dei contratti pubblici, che, seppure aggiornato e integrato nel 2016, presenta notevoli difficoltà attuative. Questo per dire che il disegno di legge delega che discutiamo, approvato dal Governo nel giugno 2021, rientra proprio nelle riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e intende, al fine di evitare procedure di infrazione, certamente recepire le tre direttive UE (la 24 e la n. 25 del 2014), in merito alla riduzione e alla certezza dei tempi relativi alle procedure di gara, alla stipula dei contratti, alla realizzazione di opere pubbliche, alla digitalizzazione e informatizzazione delle procedure, alla semplificazione e all'ampliamento delle forme di partenariato pubblico-privato. in esame vuole ridurre al massimo le regole che vanno oltre quelle richieste dalla normativa europea, comparando invece la normativa italiana con quella adottata anche in altri Stati membri dell'Unione, soprattutto tenendo conto delle discipline normative dei Paesi che da tempo attuano in modo concreto la semplificazione e la velocizzazione delle procedure. In Commissione lavori pubblici e comunicazioni qui in Senato abbiamo discusso molto sul testo di questo disegno di legge e di ciò ringrazio il Governo, nelle persone del vice ministro Bellanova e del ministro D'Incà, e i relatori, senatori Pergreffi e Cioffi. Forza Italia, che ha sempre condiviso la riforma del codice, ha dato il suo contributo con la proposta di diversi emendamenti migliorativi del testo, anche sulla base dell'audizione di soggetti interessati, ossia quelle persone e quelle aziende che quotidianamente affrontano la difficoltà di applicazione nel concreto della normativa e le lungaggini burocratiche. Con i colleghi tutti, anche con quelli dell'opposizione, che ringrazio in modo particolare per il contributo che hanno dato per far andare avanti i lavori in modo più sereno,

dei relatori, ma che rappresenta un punto di inizio per risolvere le criticità presenti nell'attuale codice degli appalti, il quale, prima di contenuti veri e propri, manca di chiarezza e semplicità espositiva. espositiva. Successivamente all'approvazione della legge, i decreti attuativi saranno adottati entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, a cura del Consiglio di Stato. Su quanto stabilito dalla legge e voluto in questo caso fortemente dal Governo non mi soffermo, pur condividendo le perplessità evidenziate *in primis* dai relatori, ma anche dal collega Paroli in modo chiaro. Bisogna che questi decreti attuativi prevedano quindi una maggiore chiarezza di linguaggio e, per quanto riguarda il merito, assicurino il rispetto dei criteri espressi dal Parlamento: con una semplificazione della disciplina applicabile a tali settori, e tenendo conto anche delle specificità. Questo è proprio frutto di un emendamento di Forza Italia, condiviso con tutte le forze di maggioranza, nel settore dei contratti nell'ambito dei beni culturali, con la previsione del divieto per le stazioni appaltanti di utilizzare, ai fini della selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazione particolari e specificamente motivate. la ridefinizione della disciplina in materia di stazioni appaltanti, con un potenziamento e un'attenzione particolare per la formazione e specializzazione del personale, oltre alla prospettiva di una stabilizzazione del personale precario, regolamentando in modo adeguato anche il *turnover.* Bisogna pensare alla riduzione dei tempi di realizzazione delle opere pubbliche, con interventi puntuali sulle procedure relative alla fase di approvazione dei progetti, anche ridefinendo e riducendo i livelli di progettazione e snellendo le procedure di verifica e validazione dei progetti e favorire poi, attraverso misure reali, gli investimenti in tecnologie *green* e digitali per rientrare negli obiettivi dello sviluppo sostenibile, del rispetto di responsabilità ambientale ed energetica. Questi sono solo alcuni *flash.* Gli argomenti cardine di questa legge delega sono i soliti, sono quelli più antichi che da tempo richiedono risposte e che oggi però abbiamo la possibilità concreta di riprendere, di attualizzare e di contestualizzare, per consentire effettivamente la realizzazione di quella riforma che aspettavamo da tempo e per cui è necessario soddisfare le attese con un impegno tangibile del Governo in piena collaborazione con il Parlamento sia per l'incidenza storica del PIL degli acquisti pubblici, pari a circa l'11 sia per le significative prospettive di spesa e investimento abilitate dal PNRR, per rendere utilizzabile quindi ogni strumento a disposizione prima che sia troppo tardi. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero innanzitutto rivolgere un ringraziamento veramente sentito alla Vice Ministro, ai due relatori e alla Commissione tutta, compresa la minoranza, per il lavoro che è stato svolto, effettivamente

ormai le norme europee non consentivano più di andare avanti con il vecchio codice, eravamo in alcuni casi in infrazione e quindi si doveva andare a porre rimedio andando a definire grazie a tutti

A questo punto, non possiamo però permettere che questa esperienza, questo successo resti semplicemente una parentesi: bisogna prendere esempio da ciò che si è fatto di buono e portarlo avanti. Nei contenuti, serviva quindi dare una delega al Governo perché venisse definito un codice più aderente alle norme europee, che non prevedesse delle

Serve una riduzione dei tempi, avere una certezza dei tempi per fare questi lavori. Serve snellire le procedure, velocizzare le risposte che vengono date al mondo del lavoro,

quelle a chilometro zero. Questo attraverso l'impedimento di suddivisione in lotti fittizi o l'accorpamento di lotti fittizi.

perché anche qui bisogna andare su ciò che si conosce e che funziona. Sono stati definiti criteri ambientali minimi: è giusto; siamo in un

un altro tassello del PNRR dovrebbe andare a posizione. Un altro tassello che questa volta mi aveva colto con un po' di fiducia in più rispetto alla consueta attività del Governo. Quando il mio collega e capogruppo in Commissione, senatore Ruspandini, mi ha comunicato infatti che questa volta non venina posta la fiducia, ho pensato che finalmente le parole del presidente Mattarella e - ci sia permesso citare con molta minore importanza - le richieste reiterate dell'opposizione per un maggior coinvolgimento del Parlamento avessero avuto effetto. Nella fattispecie lo hanno avuto; ciò ci fa piacere e speriamo che sia di buon auspicio per il prosieguo dell'attività legislativa e parlamentare.

raramente abbiano visto un Parlamento delegare il Governo e poi, a sua volta, il Governo delegare di fatto un altro organo dello Stato a svolgere le proprie funzioni. Quando poi verifichiamo nella fattispecie, con la massima stima e rispetto per il Consiglio di Stato, che questa delega viene data ad un organo giurisdizionale, chi un po' ne capisce di procedure, atti amministrativi, appalti, bandi e gare, qualche problema se lo pone sia da un punto di vista politico e democratico, perché l'eccesso di delega non è mai positivo,

l'esecutività dei lavori, il fatto che davvero si possa poi trasformare in opere concrete quanto il PNRR

a un organo giurisdizionale la funzione di delega. Si poteva invece condividere un percorso dove il Governo, mantenendo comunque la regia e il ruolo, condividesse con dei tecnici giurisdizionali, ma anche dell'impresa e del privato, questo *iter*. Per tale motivo la mia analisi

e in più a una delega in bianco che è una doppia delega con l'intervento del Consiglio di Stato. Signor Ministro, mi permetta, come opposizione che non vuole certamente precostituire critiche, ma cercare di portare un contributo di proposizione e di miglioramento,

Nel merito del provvedimento, mi sia permesso di fare riferimento ad un passaggio che abbiamo sicuramente condiviso. Mi riferisco al divieto di unire i lotti; questione che di fatto ha spesso precluso

concreta delle opere che i vari bandi e appalti devono poi garantire. Avremmo avuto piacere che la maggioranza fosse più aperta al ruolo dell'opposizione, fosse più aperta alle proposte che l'opposizione, sempre con quella serietà che vorremmo potesse contraddistinguerci, ha esercitato in sede di Commissione.

che avevano qualche problema con il DURC o irregolarità fiscale non definitiva. Infatti, ricordiamoci sempre - lo dico da commercialista - che gli accertamenti dell'Agenzia delle entrate sono non un mantra, bensì il parere di una parte che dovrà essere eventualmente accettato con il pagamento dal contribuente, ovvero contestato e giudicato dagli organi giudicanti. Pertanto, finché l'atto di accertamento non diviene definitivo,

è dovuta a una irregolarità dello Stato, delle Regioni, dei Comuni e di tutte quelle pubbliche amministrazioni che non le hanno pagate. Signor Ministro, capirà che accogliere quell'emendamento di Fratelli d'Italia sarebbe stato un atto di giustizia verso il sistema Italia e non un favore a una forza di opposizione.

anche lì vediamo che il Governo vuole mantenere il controllo assoluto per poter poi - dobbiamo dircelo e dirlo ai cittadini e agli elettori che ci ascoltano - legiferare tramite i decreti delegati

Nell'ambito della riforma tributaria, un tema che sta facendo parlare tanti e arrabbiare molti è la riforma del catasto. non si può però dire agli italiani che si fa la riforma del catasto, ma non si aumentano le tasse. Forse non si aumenteranno domani, ma se si fa la riforma del catasto - lo capisce anche un ragazzino della quinta elementare - prima o poi (purtroppo più prima, che poi) le tasse verranno ulteriormente aumentate.

Andremo a penalizzare ancora di più quei risparmiatori italiani che hanno cercato con tutte le loro forze di risparmiare e, invece di essere premiati, vengono disincentivati con maggiori tassazioni. Non risolviamo così i problemi, peraltro in un momento nel quale le casse dello Stato sono già in difficoltà e lo sono ancora di più quelle dei cittadini a causa della crisi energetica che li sta colpendo in modo brutale.

Credo di non essere l'unico in quest'Aula a ricevere giornalmente grida di dolore da povera gente che vorrebbe pagare i propri debiti con lo Stato. Mi riferisco alle cartelle esattoriali rottamazione-*ter* e saldo e stralcio. Questi cittadini vorrebbero pagare, ma lo scorso anno,

Parliamo di un mercato che solo nel primo quadrimestre 2021 ha generato un volume di circa 70 miliardi di euro, considerando tutte le tipologie. Il disegno di legge delega in materia di contratti pubblici è stato messo a punto al fine di assicurare un riordino e una rivisitazione complessiva del codice degli appalti, rispetto al quale nel corso degli anni sono stati introdotti numerosi cambiamenti, anche attraverso provvedimenti d'urgenza, che hanno profondamente modificato l'originario impianto del codice stesso. Come è noto, la normativa dei contratti pubblici ha subito nel corso degli anni numerosi interventi correttivi, integrativi, modificativi, derogatori che, seppure a volte necessari, in molti casi non hanno aiutato il settore; interventi che hanno finito per rendere l'intero impianto normativo disordinato, troppo complicato per tutti gli operatori pubblici e privati. Sappiamo tutti quanto sia di fondamentale importanza il principio di affidamento nel nostro ordinamento, che in questa materia che interviene sui settori chiave e strategici, rappresentando un volano di notevolissimo impatto per l'intera economia nazionale, la certezza del diritto rappresenta un principio irrinunciabile. Oggi, alla luce delle risorse destinate all'Italia dal PNRR, l'ambito degli appalti acquisisce un'importanza ancora maggiore e noi siamo chiamati ad approvare una disciplina la più chiara possibile, soprattutto di agevole applicazione per tutti gli operatori, se crediamo veramente nella ripresa della nostra economia. Abbiamo davanti un calendario molto stringente e questa riforma rientra, tra l'altro, tra gli impegni precedentemente assunti dal Governo per il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Nello stesso piano, infatti, si prevede una riforma complessiva del quadro legislativo nel settore dei contratti pubblici e, in base a quanto previsto, devono essere raggiungi obiettivi in tempi molto rigorosi: alla fine del prossimo anno il quadro normativo e attuativo deve andare in porto definitivamente, non possiamo permetterci ritardi o esitazioni e per questo auspico un passaggio alla Camera che, pur rispettoso del confronto tra le varie forze politiche, resti dentro limiti di tempo non lunghi. Questo lo voglio dire anche perché non è escluso che una parte della crescita economica prevista per il nostro Paese grazie alle risorse messe in moto dal *recovery plan* venga vanificata dagli effetti nefasti della guerra in Ucraina. Il disegno di legge delega si configura come un intervento normativo volto ad adeguare la disciplina dei contratti pubblici a quella del diritto europeo e ai principi espressi nel corso degli anni dalla giurisprudenza in tale materia, il cui obiettivo complessivo è quello di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente. Gli assi portanti del disegno di legge governativo messi in risalto nei principi e criteri direttivi della delega sono riassumibili nel divieto di *gold plating* che, in linea con le direttive europee, impedisce l'inserimento nella normativa nazionale di livelli di regolazione maggiori rispetto a quelli minimi previsti, nella qualificazione delle stazioni appaltanti. Il disegno di legge delega, infatti, stabilisce chiaramente che uno degli obiettivi è quello di conseguire una riduzione numerica, favorire un accorpamento di quelle esistenti, promuovere incentivi finalizzati all'utilizzo delle centrali uniche di committenza e potenziare la qualificazione del personale. In questa direzione va un nostro emendamento, con il quale si invita a procedere ad una razionalizzazione delle stazioni appaltanti, con riferimento sia a quelle afferenti ai settori ordinari che a quelle afferenti ai settori speciali.

e questo, come dicevo, non aiuta gli operatori del settore e le pubbliche amministrazioni che, al contrario, hanno bisogno di regole chiare e durature. Si interviene altresì nella normativa relativa ad investimenti in tecnologie verdi e digitali. In questo ambito sarà importante procedere con un vero e proprio disegno strategico, finalizzato alla semplificazione delle procedure, in modo da realizzare, in linea con le due transizioni previste, gli investimenti *green* e digitali. L'emendamento del senatore Margiotta, approvato in Commissione, è inteso a estendere e rafforzare l'ecosostenibilità degli investimenti pubblici, con l'inserimento del principio della rendicontazione degli obiettivi energetico-ambientali. Si vuole quindi garantire non solo la fase a monte della definizione dei criteri, ma anche la fase a valle della rendicontazione dei risultati raggiunti in termini di sostenibilità ambientale ed energetica. In chiave di informatizzazione delle procedure per ridurre i tempi relativi alle procedure di gara, di stipula dei contratti e di esecuzione dei lavori, grazie a una modifica del disegno di legge, si stabilisce, anche al fine di evitare ulteriori gravami a carico degli operatori economici, il divieto di addebito agli operatori economici di qualsiasi tipologia di costo, anche indiretto, connesso alla gestione di piattaforme elettroniche. Il disegno di legge delega si estende anche su altri ambiti, sui quali, per ragioni di tempo, non mi soffermerò. Ci tengo, però, a dedicare qualche considerazione al lavoro svolto in Commissione e mi sia consentito un ringraziamento sincero ai relatori, la collega Pergreffi e il collega Cioffi, oltre che ai colleghi del Partito Democratico, a partire dal capogruppo Margiotta, e a tutte le forze politiche nella Commissione. Il lavoro in Commissione è stato molto intenso e impegnativo, i tempi di esame si sono allungati per via della necessità di trovare la più ampia convergenza, specie sui passaggi più delicati del provvedimento, oltre che per la complessità della materia, che richiede inevitabilmente margini di riflessione più lunghi. Tuttavia, anche dal confronto con il Governo (e voglio rivolgere al vice ministro Bellanova un ringraziamento sincero e non di forma, perché ha lavorato in maniera preziosa con le forze parlamentari), possiamo dire che il testo arrivato in Assemblea risulta migliorato in più punti e ne vorrei ricordare qualcuno. Tra questi, certamente rientrano gli emendamenti finalizzati a sancire il principio della inderogabilità delle misure a tutela del lavoro, della sicurezza e del contrasto al lavoro irregolare, della legalità e della trasparenza. La tutela del lavoro e la sicurezza dei luoghi di lavoro è un tema che impone a tutti noi la massima attenzione, sempre, non soltanto davanti agli incidenti o alle morti sul lavoro. Oggi, alla luce dei numerosi *bonus* edilizi, che nel loro complesso stanno funzionando bene, l'impianto attuativo di tale principio deve essere stringente e molto rigoroso. Non possiamo dimenticare, a un mese e mezzo di distanza, l'ammonimento del presidente Mattarella nel giorno del suo giuramento, quando ci ha sollecitato ad «azzerare le morti che feriscono la società e la coscienza di ognuno di noi. Perché la sicurezza del lavoro, di ogni lavoratore, riguarda il valore che attribuiamo alla vita». Dello stesso tenore, perché tocca il tema della sicurezza e dei suoi costi, è l'emendamento in cui si prevede che i costi della manodopera e della sicurezza siano sempre scorporati dagli importi assoggettati a ribasso. Alla luce del fenomeno al quale stiamo assistendo, relativo al notevole aumento dei prezzi nel settore dei lavori pubblici, l'emendamento che abbiamo proposto e approvato, finalizzato a prevedere un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di condizioni di oggettiva eccezionalità e imprevedibilità al momento della formazione dell'offerta, coglie un punto di stretta attualità e, anche per il futuro, rappresenta un presidio di notevole importanza nei casi in cui si verificassero aumenti consistenti delle materie prime. Vi è poi il principio della inderogabilità del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, quindi il divieto del massimo ribasso, che è stato inserito - ritengo giustamente - nei contratti pubblici relativi ai servizi sociali e della ristorazione ospedaliera, dell'assistenza scolastica, nonché a quelli del servizio ad alta intensità di manodopera, dove è evidente che tale criterio è quello che offre migliori garanzie circa il buon esito dell'affidamento, soprattutto in settori sensibili. Per concludere, quindi, con l'approvazione di questo provvedimento andiamo a migliorare alcuni fondamentali punti di questa materia: dalla semplificazione di norme e procedure, al rispetto per l'ambiente, allo stop ai massimi ribassi in alcuni settori, agendo sui costi del lavoro e della sicurezza e ponendo attenzione al sociale e all'obbligo di revisione dei prezzi da parte delle stazioni appaltanti. È un testo centrale, questo, per l'attuazione del PNRR e per la ripartenza del nostro Paese.

Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame, la delega al Governo in materia di contratti pubblici, ha avuto un proficuo *iter* in 8a Commissione. Basti pensare che consta di un solo articolo, sul quale sono stati presentati qualche centinaia di emendamenti. Grazie all'apporto di tutte le componenti politiche, il testo è stato licenziato celermente, ma con modifiche decisamente mirate, migliorandolo e mantenendo salde le finalità del provvedimento ovvero semplificare, razionalizzare, riordinare la disciplina e, su tutto, evitare l'avvio di procedure di infrazione. I principi e i criteri direttivi, che il provvedimento individua e ai quali il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega, sono: la semplificazione della disciplina, che sarà così applicabile a tutti quei contratti pubblici che vedono lavori, servizi e forniture inferiori alle soglie di rilevanza europea. Importantissimo è il passo in avanti fatto per il conseguimento degli obiettivi dell'Agenda 2030,

La razionalizzazione, limando tutte quelle farraginose storture che prima ingolfavano i procedimenti, e l'avanzare delle pratiche porteranno comunque vantaggi, che si avranno con la riduzione e la certezza dei tempi relativi alle procedure di gara, alla stipula dei contratti e all'esecuzione degli appalti. L'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara avvisi di inviti specifiche clausole sociali non può che essere una scelta di buon senso; saranno fondamentali per la promozione e la stabilità occupazionale del personale impiegato, per garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, per promuovere le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità. L'obiettivo primario era di migliorare, talvolta sradicare, il codice degli appalti approvato nella scorsa legislatura, che era forse troppo fedele alle tre direttive comunitarie alle quali faceva riferimento e poco adatto alle peculiarità italiane. Ha difatti talvolta disorientato, viste le abitudini e i tempi di reazione legislativa del nostro Paese, ed è stata la stessa Autorità garante per la concorrenza che ci ha indotti a imprimere questo cambio di passo. La disciplina del codice dei contratti pubblici è stata negli anni stigmatizzata per la complessità, aggravata dai numerosi e troppo spesso inconcludenti rinvii a futuri provvedimenti attuativi. Prima le linee guida Anac poi è stata la volta del noto regolamento attuativo introdotto dal cosiddetto sblocca cantieri. Questi provvedimenti hanno privato gli operatori della consegna di una disciplina certa e coordinata e trasformato la gestione dell'attuale codice in una lunga attesa di decantazione normativa, che si è protratta troppo a lungo nel tempo, non dando spazio a quella celerità e a quella certezza della burocrazia che aiutano ad attivare la macchina economica del Paese ovvero le difficoltà incontrate da stazioni appaltanti e operatori economici con l'applicazione della normativa in vigore fino ad oggi, prima del provvedimento che stiamo discutendo. Nel ringraziare il Presidente della Commissione, i relatori, il Governo e i colleghi di tutte le forze politiche, rilevo che è stato davvero un lavoro di squadra, straordinario esempio di un Parlamento che, *in primis*, guarda alla cosa pubblica. Mi preme sottolineare l'importanza di aver dato il giusto spazio ad ognuno di noi, consentendo a ciascuno di apportare il proprio contributo. Si dice che non esistono leggi perfette, ma noi consegniamo al Governo un buon lavoro. Era quanto si aspettavano le imprese italiane per un nuovo percorso. Nel dettaglio, con l'approvazione dei nostri emendamenti abbiamo premuto per la revisione dei prezzi obbligatoria, l'adozione di un regolamento attuativo in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, la razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclusione, al fine di rendere le regole di partecipazione chiare e certe, individuando le fattispecie che configurano l'illecito professionale; ancora, la semplificazione delle procedure di pagamento da parte delle stazioni appaltanti del corrispettivo contrattuale, anche riducendo gli oneri amministrativi a carico delle imprese. Abbiamo scandito i tempi di attuazione dei decreti attuativi, ma soprattutto abbiamo posto attenzione alle piccole e medie imprese. Sono stati tempi difficili per l'economia di questo Paese. Il benessere dei cittadini passa attraverso la creazione del lavoro. Ebbene, per una ripresa davvero valida era necessaria la semplificazione delle procedure di acquisto, che tra l'altro costituisce un obiettivo del PNRR ai fini di un'efficiente realizzazione delle infrastrutture per il rilancio dell'attività edilizia, entrambi aspetti essenziali per la ripresa a seguito della diffusione del contagio da Covid-19. La ripresa economica viene minata purtroppo ancor più oggi dalla situazione economica più oggi dalla situazione economica aggravata dalla crisi Ucraina e dal caro energia di materie prime che ne deriva. Come Commissione e come Parlamento abbiamo lavorato rapidamente e con buon senso per non sprecare questo momento favorevole che vede l'incidenza storica sul PIL degli acquisti pubblici pari a circa l'11 per cento, come riportato anche dall' Autorità garante della concorrenza e del mercato, e per consolidare e aumentare le significative prospettive di spesa e investimento consentite dal PNRR. Oggi, per far sì che tali aspettative vengano soddisfatte, il Parlamento consegna all'Esecutivo un ottimo strumento. Noi, come componente, accogliamo positivamente questo provvedimento e siamo sicuri che verrà adottato in tempi certi e rapidi - naturalmente quelli che il Parlamento ha assegnato - e siamo altresì consapevoli che costituirà un punto qualificante di riforma per un settore che nutre notevole aspettative.

Governo, colleghi, parto da una premessa che è fuori tema. Apprendo da conoscenti che il gasolio alla pompa oggi ha raggiunto 2,4 euro; apprendo che l'acciaio e il ferro non vengono consegnati a nessun prezzo e a nessuna condizione. Penso che la bomba atomica non l'abbia Putin, ma l'abbiamo noi sotto i nostri sedili, sotto le nostre sedie. Tra qualche giorno parleremo d'altro, con un'inflazione reale non controllabile, con fallimenti, disoccupazione e problemi difficili da affrontare. Lo dico per conoscenza ma in spirito di verità e di servizio. Veniamo al tema Questo dibattito resterà agli atti parlamentari e spero che il Governo ascolti e recepisca magari qualche nota degna di essere tradotta poi in normativa specifica nel decreto legislativo. Su questi temi si parte sempre dalla necessità di adeguarsi alla normativa europea, la quale obbedisce ad alcuni principi - ne parlavamo in Commissione in questi giorni - quali la concorrenza, la competitività, la tutela del consumatore. L'Italia dovrebbe suggerire che al posto di "consumatore" potremmo scrivere "cittadino"; ma la concorrenza e la competitività che cosa sono? Si può fare utile, si può lavorare sulla qualità, sul rispetto dei tempi, oppure guadagnare è peccato? È una cosa che mi arrovella sempre il cervello. Credo che bisogna obbedire a regole di concretezza e realtà. noi diamo una delega al Governo per scrivere questo decreto legislativo, che per forza di cose sarà fatto di norme concrete. Non so se la delega sia troppo generica, troppo ampia o se sia esaustiva. Ho letto delle cose interessanti, mi associo a quanto detto dai colleghi di tutti gli schieramenti. Si vuole far scrivere e chiedere l'aiuto senza corrispettivo al Consiglio di Stato o all'Avvocatura, ma mi pare che soprattutto il Consiglio di Stato sia il controllore, non sia il regolatore.

sono già stati stanziati 130 milioni con un primo decreto per il 2021; 100 milioni nella legge di bilancio (commi 398 398 e 399); 150 milioni nel decreto-legge n. 17. Sono cifre importanti, ma rispetto all'aumento dei prezzi su qualche decina di miliardi di appalti potenziali nel 2022,

alla tipizzazione dei casi per il criterio del massimo ribasso, quest'ultimo è pericoloso perché può attirare l'interesse di ditte costituite all'uopo, che poi una volta vinto l'appalto si eclissano o cominciano con le eccezioni. limitata a casi assolutamente minori, altrimenti non è il metodo giusto. Le procedure flessibili, che sono state citate e recepite, sono buone perché consentono alle stazioni appaltanti di risolvere i piccoli problemi,

grazie a tutti

riduzione dei livelli di progettazione e validazione, si potrebbe scrivere una casistica per cui in certi casi il definitivo e l'esecutivo può essere un unico passaggio.

pagamento degli acconti, quando si eseguono lavori pubblici sulla base di contributi dallo Stato o dalle Regioni ad enti inferiori, si presenta un problema di cassa, perché giustamente bisogna pagare l'anticipo

Bisogna razionalizzare il controllo sugli investimenti e sulla loro quantificazione, ai fini della concessione per la restituzione da parte del subentrante e questo è un argomento delicato che andrebbe previsto prima in maniera che il il computo degli investimenti sia fatto secondo i prezzi vigenti o secondo criteri stabiliti. Le sanzioni, in caso di errore o disattesi le aspettative e gli obblighi contrattuali, siano proporzionate all'inadempimento e comminate in tempi rapidi, con provvisoria esecutività delle revoche, altrimenti dopo che ne veniamo fuori si innescano meccanismi di interpretazione, che sono sempre a danno dello Stato.

Sei mesi di tempo per l'adozione dei decreti legislativi sono pochi da un lato, ma con quello che sta succedendo in questi giorni sono un'eternità. Auspichiamo che siano ridotti al minimo. Confido nella parte migliore della pubblica amministrazione - che c'è - e in questi suggerimenti alla luce del presente dibattito.

Colleghi, non deve essere certamente la procedura di infrazione da parte della Commissione europea a imporci la revisione della disciplina dei contratti pubblici, ma il buon senso della politica e soprattutto il rispetto del lavoro delle imprese italiane. La lega ha cuore i lavori e tutta la macchina amministrativa ad essi legata, e la prova ne sono gli emendamenti presentati e anche approvati, i quali promuovono un cambio di passo con una riorganizzazione del settore più più tempestiva e organica, a partire anzitutto dalla normativa. Il testo licenziato dalla Commissione getta le basi per una nuova legge sui contratti pubblici più snella e anche maggiormente equilibrata. La Lega ha arricchito la legge delega con una serie di emendamenti che hanno come principio il rispetto del sacrificio e del rischio dell'impresa. Penso, ad esempio, all'emendamento per la tutela del *made in Italy* nelle forniture, all'emendamento per il ravvedimento dei costi in caso di aumenti controllati (vedasi oggi l'aumento delle materie prime e del costo dell'energia). Penso ancora all'emendamento che dà la possibilità anche alle piccole imprese di partecipare a grandi appalti perché spartiti in piccoli lotti. La Lega fa così crescere le piccole imprese territoriali e velocizza il lavoro delle grandi. Gli emendamenti della Lega prevedono la semplificazione delle regole che configurano l'illecito professionale e l'individuazione delle cause vere che determinano l'esclusione dai bandi, perciò risposte chiare e concrete di sostegno. Tutto ciò non solo per una disciplina in linea con le direttive già da tempo richieste o per il conseguimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, ma soprattutto per fare in modo di poter organizzare le attività ad investimenti materiali e amministrativi. Gli emendamenti proposti sono finalizzati a incentivare una buona e celere esecuzione dei lavori anche mediante meccanismi sanzionatori o premiali. Occorrono infatti regole che scongiurino opere incompiute, come le 410 opere al 2020 dal valore di oltre 2,5 miliardi. Al riguardo, nelle more anche di un rapido controllo e monitoraggio, ben venga l'ordine del giorno della Lega che promuove la digitalizzazione del settore italiano delle costruzioni e delle pubbliche amministrazioni. La Lega ha presentato e strutturato nella delega al Governo un emendamento per limitare il ricorso al sorteggio, perché crediamo sia giusto premiare la professionalità. Con l'emendamento 1.155 abbiamo voluto che si prevedessero prevedessero polizze assicurative a carico della stazione appaltante. Con l'ordine del giorno (già emendamento 1.81) riconosciamo il ruolo determinante dei professionisti coinvolti nella partecipazione a gare. Con l'emendamento 1.247 (testo 2) interveniamo nel valore oggettivo e sociale del servizio di ristorazione collettiva. In esso ha valore nutrire ed educare bambini, anziani e malati e si premia la qualità dell'offerta con criteri che valorizzano le politiche di approvvigionamento alimentare e si raccomandano criteri che premiano la progettualità di comunicazione e informazione, con una prevenzione degli sprechi e una sostenibilità dei pasti, si verifica altresì l'affidabilità socio-economica e le certificazioni e si determina inoltre l'esclusione dagli appalti della ristorazione collettiva di una ristorazione improvvisata. Abbiamo strutturato l'emendamento che valorizza l'esperienza professionale maturata negli anni dai direttori tecnici, dando ancora una volta priorità alla meritocrazia e alla professionalità. Il lavoro della e nella Commissione, a cui va il ringraziamento per il proficuo e costruttivo impegno, a cominciare dagli uffici, dai colleghi, dai relatori, in modo particolare la senatrice Pergreffi, e dal Governo, con la presenza costante e costruttiva della senatrice vice ministro Bellanova, spero trovi effettiva delega al Governo perché l'impegno profuso ha strutturato una serie di emendamenti che creeranno sintesi per buone regole dei contratti pubblici. Come anche per tale legge delega, la Lega è al Governo per il bene delle imprese e dei suoi professionisti. Se non fossimo al Governo, avremmo solo ipotizzato, senza portare a complimento idee e richieste in grado di dare risposte, certezze e programmazione. Per la Lega è il momento di essere anche criticati, ma non di criticare; è il momento di fare, ma non di lasciar fare. Per il bene degli italiani ci mettiamo sempre la faccia. la delega che stiamo conferendo oggi al Governo rappresenta il superamento di uno scoglio sul quale ripetutamente si sono abbattute stazioni appaltanti ed operazioni del settore, ma non per la grave emergenza economica e sanitaria in cui anche il nostro Paese si è trovato a navigare. Solo in questa legislatura si sono rese necessarie numerose modifiche al codice degli appalti. Ne ricordo solo alcune: il decreto cura Italia, il decreto rilancio, il decreto semplificazioni del 2020 e quello del 2021. Sono stati tutti interventi necessari, ma non sufficienti. È rimasta ad esempio la viva necessità di adeguamento della normativa al diritto europeo sia per permettere di giungere alla risoluzione di procedure di infrazione già avviate sia per evitarne l'avvio di nuove. Ciò soprattutto perché da sempre da parte degli operatori economici c'è la richiesta di razionalizzare, riordinare e semplificare una disciplina che

le problematiche applicative legate alla sua stessa entrata in vigore, che rappresentano lo scoglio sul quale gli operatori del settore tornano e ritornano ad infrangersi. Un quadro giuridico poco chiaro e poco organico, soggetto a perenni modifiche puntuali che con l'emergenza da Covid-19 si sono acuite e con le quali si è derogato al fine di semplificare l'approccio per la gestione della fase pandemica. In Commissione è approdato un testo dal quale si è immediatamente evinto il fine primario: restituire alle disposizioni codicistiche un linguaggio semplice e chiaro, limitando il più possibile il rinvio a norme secondarie, prevedendo una riforma complessiva del quadro legislativo in materia di contratti pubblici e rispettando l'impegno recentemente assunto dal Governo con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, che prevede l'entrata in vigore della delega per la revisione del codice dei contratti pubblici entro il mese di giugno 2022. *(Applausi)*. Oggi, 9 marzo 2022, posso dire che nonostante il contingentamento dei tempi, il dibattito è stato molto alto tra il Parlamento e il Governo. Voglio anzitutto ringraziare tutti i colleghi di Commissione per gli importanti momenti di condivisione e di illustrazione delle proprie idee, a volte anche divergenti, sulle quali siamo riusciti però a trovare una sintesi. Voglio ringraziare anche il Governo che, con la sua apertura su vari fronti, ha permesso al Parlamento di contribuire in maniera significativa al miglioramento del testo, che delinea una cornice entro la quale muoversi per riformare la materia del codice dei contratti pubblici. *(Applausi)*. Una buona base di partenza, ad esempio, era già indicata nell'articolo 1, alla lettera c, sulle semplificazioni delle procedure finalizzate alla realizzazione di interventi in tecnologie verdi, digitali, di innovazione e di ricerca. Facendo esplicito riferimento alla necessità del perseguimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, l'azione del Parlamento ha saputo introdursi ponendo l'accento sull'obbligatorietà del rispetto dei criteri minimi ambientali. Infatti, se già la delega mostrava l'importanza dell'uso e della leva di questi criteri, l'inserimento della previsione dell'obbligo fa intendere quanto questo strumento abbia la possibilità di cambiare il nostro Paese. Inoltre, abbiamo introdotto la rendicontazione degli obiettivi energetico-ambientali, ovvero quel sistema che consente di misurare l'effettivo impatto necessario al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030, esattamente come da deliberazione del 2015 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

ambientale nell'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione. Tra le tante, una delle tematiche più fortemente partecipata da tutti i Gruppi parlamentari è stata certamente quella che tutela, preserva e favorisce la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese agli appalti pubblici. Occorre qui partire da un dato di fatto: per cento delle imprese italiane ha un numero di addetti ricompresi tra le nove e la singola unità. In tutta onestà, possiamo quindi asserire che la quasi totalità del mercato è composta da micro, piccole e medie imprese. Il testo di delega non prevedeva alcuna menzione di questa tipologia di imprese, che di fatto rappresenta l'ossatura produttiva del nostro Paese. La discussione in Commissione ci ha trovato tutti coerentemente concordi nel mettere a punto un principio di delega che ne definisse la tutela, al fine di garantire loro l'effettiva possibilità di partecipare alle gare, prevedendo un'adeguata suddivisione dei lotti sulla base qualitativa e quantitativa e impedendone l'accorpamento artificioso. Signor Presidente, in questo modo andiamo davvero a tutelare il mercato italiano e le imprese che maggiormente lo rappresentano. Certezza dei tempi: si tratta dell'annosa tematica affrontata nel testo, ma decisamente migliorata grazie all'approvazione di un emendamento proposto dal MoVimento 5 Stelle, che mira a introdurre nel criterio di delega il riferimento alla piena attuazione della banca dati nazionale dei contratti pubblici e l'utilizzo del fascicolo virtuale dell'operatore economico, innalzandoli a elementi cardine del processo di semplificazione delle procedure di gara. Il fascicolo elettronico è uno strumento che - a oggi - non viene ancora usato al pieno delle sue potenzialità, mentre il MoVimento 5 Stelle ritiene fortemente che questa puntuale modifica emendativa nel dettaglio possa davvero contribuire al raggiungimento di tale obiettivo. La delega prevede, inoltre, un criterio volto a specificare le procedure relative alla fase di approvazione di progetti anche attraverso un'eventuale riduzione dei livelli di progettazione e la razionalizzazione dell'attività e della composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Ebbene, c'è da dire che la normativa che interviene nell'*iter* di approvazione, affidamento e realizzazione delle opere pubbliche è particolarmente articolata in molte occasioni contempla una pluralità di fonti, come codice dell'ambiente e codice dei beni culturali e del paesaggio. Questo incastro di norme comporta una complessa opera di raccordo tra disposizioni assai articolate. In tal senso, tutti i Gruppi parlamentari si sono mostrati sensibili e, sebbene da un chiaro confronto con il Governo sia venuto alla luce che non era esattamente questo il provvedimento adatto a intervenire per un coordinamento tra questi testi, tutte le forze politiche dell'arco parlamentare, opposizione inclusa, si sono unite nella formulazione di un ordine del giorno, promosso dal MoVimento 5 Stelle e accolto dal Governo, che invita, in sede di adozione dei decreti legislativi, a garantire il coordinamento tra il codice dell'ambiente, il codice dei beni culturali e del paesaggio, il codice dei contratti pubblici e tutte le altre eventuali discipline interessate. conclusione, ritengo che il lavoro svolto in Commissione e che ora ci apprestiamo a votare in quest'Aula sia stato svolto in maniera corale e coinvolgente. Nel ringraziare soprattutto entrambi entrambi i relatori per il prezioso e paziente lavoro di mediazione svolto, mi auguro sinceramente che questa modalità possa essere adottata anche per il prosieguo dei lavori. *(Applausi)*.

questo è uno scopo interessante che si era proposto la Commissione, come avevamo già detto, in ossequio alla modifica costituzionale, che è uno dei risultati raggiunti in maniera corale da tutte le forze parlamentari. Il senatore Astorre parlava della riduzione delle stazioni appaltanti: anche questo è un grande tema. Sappiamo che all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) sono iscritte 37.000 stazioni appaltanti, un numero sicuramente incredibile,

è assolutamente necessaria e spero che il Governo ci lavori con attenzione, ovviamente in accordo con la Conferenza Stato-Regioni, per trovare un equilibrio.

dovrà stare particolarmente attento a non intervenire con continue modifiche che determinano quell'incertezza normativa che produce un vero problema nell'attuazione dei lavori.

In ultimo, molti rappresentanti di tutte le forze politiche hanno fatto riferimento al Consiglio di Stato (il senatore Paroli, la senatrice Lupo, il senatore Corti, la senatrice Vono,

Se volessi fare una battuta, potremmo dire scherzosamente che il Governo dei migliori ha scelto qualcuno migliore di loro per farsi migliorare. Questa rimane una battuta, ma il problema, a volte, è che alcune alcune componenti giuridiche e alcuni funzionari giuridici si sentono, come gli x-men, in grado di salvare il mondo. Noi pensiamo invece che la politica debba essere al centro, come ripetiamo sempre in queste Aule parlamentari. Dobbiamo fare in modo che la separazione delle funzioni sia viva, forte ed efficace, perché, se il Consiglio di Stato scrive il decreto legislativo e qualcuno fa ricorso al Consiglio di Stato, immagino che sia difficile che il Consiglio di Stato stesso possa accettarlo, ma questa è la procedura. nella delega è scritto «ove intenda avvalersi», il nostro auspicio è che il Governo non intenda avvalersene; questo in ossequio a tutto quello che è stato detto dalle forze parlamentari, su cui c'è una grande convergenza. Il lavoro comunque è stato utile, non perfetto, come sempre succede nei lavori, ma molto efficace. Ci auguriamo che l'attuazione della delega sia ben fatta

gli Uffici della Commissione e quelli dell'Assemblea, non solo per la collaborazione, ma soprattutto per la professionalità, l'impegno e, in alcuni passaggi, direi anche la passione che ci hanno messo per approvare in Commissione un testo importante e impegnativo. Sappiamo tutti, infatti, che arriva in Aula

Arriva in Aula un testo che manderemo alla Camera, dove credo continueremo a lavorare sempre con questo approccio, sapendo che la presente delega ha una parola chiave: semplificazione; una parola tante volte evocata nel corso degli anni, ma anche tante volte assolutamente ignorata.

se non un chiarimento che, anziché avvalersi del suo parere, si potrà chiamare il Consiglio di Stato a svolgere il ruolo che gli è proprio, in base alle leggi già esistenti. Con questa delega rafforziamo quel quadro di riforme fondamentali non solo per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma anche per presidiare e sostenere la necessaria ripresa economica di cui il nostro Paese ha bisogno dopo la pandemia. Oggi diamo un contributo, attraverso il lavoro che tutti insieme abbiamo fatto, per quel patto intergenerazionale e di genere di cui sono sicura tutti in quest'Aula avvertiamo la pressante responsabilità. E questo non attiene al Governo dei migliori, ma al dovere che le classi dirigenti devono stipulare con le nuove generazioni.

il provvedimento che oggi votiamo è un importante tassello nel lungo percorso per la semplificazione del sistema. Adesso la palla passa al Governo, chiamato a mettere a terra una riforma essenziale per l'uso dei fondi europei, restituendo autonomia e sicurezza ai pubblici funzionari e alle imprese.

una riforma che, nel fare questo, deve mettere al centro il sistema imprenditoriale nella sua interezza, includendo cioè quelle piccole e medie imprese che non hanno potuto intendere il settore degli appalti pubblici come un *asset* strategico della propria attività aziendale. Tuttavia, queste imprese, che sono la dorsale economica del Paese, possono portare un valore aggiunto, non solo in termini di competenze e di professionalità, quanto di conoscenza dei territori dove si realizzano le opere. Questa prossimità, che un tempo si sarebbe chiamata sussidiarietà, è stata uno dei grandi temi al centro della discussione in Commissione. Siamo contenti che si siano apportate modifiche al testo che vanno incontro a questa esigenza. attenzione è passata da norme come quella sul divieto del sorteggio contro l'accorpamento artificioso dei lotti e quella sulla semplificazione delle procedure di pagamento. Positive in tal senso sono anche le novità legate alla revisione dei prezzi per fatti di natura oggettiva e non preventivabili, come l'introduzione di alcuni automatismi nelle valutazioni la formazione e gli interventi di sostegno per le stazioni appaltanti, che, come sappiamo, troppo spesso mancano di competenze e strumenti atti ad interpretare correttamente la propria funzione. Il secondo aspetto su cui la legge delega affida un compito molto preciso è nel cambio di passo per cui dalle mere esigenze di funzionamento del mercato si passa a un'ottica di politiche pubbliche concentrate sull'innovazione, sull'inclusione sociale e sull'ambiente. Gli esempi sono numerosi: dalle norme a tutela dei lavoratori del subappalto ai vincoli sociali sulla stabilità e l'inclusione occupazionale, al rispetto dei criteri di responsabilità energetica ambientale, alla semplificazione delle procedure per la realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali, innovazione e ricerca. In tal senso, molto importante è anche l'impegno per la semplificazione normativa del dibattito pubblico, uno strumento strategico per aiutare le amministrazioni a focalizzare punti di forza e di debolezza, rischi e opportunità di opere pubbliche ad alto impatto sui territori. Occorre incentivarne l'utilizzo abbassando l'importo economico dell'opera per cui sono obbligatori attualmente 50 milioni di euro; bisogna soprattutto sollevare da qualsiasi qualsiasi contenzioso le opere che vi hanno fatto ricorso, seguendo in questo il sistema francese. Questo perché - e qui arrivo al punto più importante - il grande tema è quello di evitare rallentamenti nella realizzazione delle opere, cosa più che mai necessaria rispetto a quelle finanziate dal PNRR, che nel 2026 dovranno essere completate. In tal senso, la legge delega stabilisce altri punti degni di nota, come il dialogo competitivo, il partenariato e le procedure competitive con negoziazione. Importante sarà poi lo snellimento delle procedure di verifica, che troppo spesso rallentano i progetti, introducendo ad esempio ancora di più il principio del silenzio-assenso nel rapporto con la pubblica amministrazione. Signor Presidente, penso si sia fatto un buon lavoro e ringrazio a questo punto *in primis* i due relatori in Commissione e il rappresentante del Governo. La Commissione, che con il Governo ha intrapreso un rapporto dialettico serrato, è riuscita ad apportare una serie di migliorie, a riprova ancora una volta dell'importanza del lavoro parlamentare nell'esame di provvedimenti così delicati e complessi. La normativa sugli appalti pubblici merita un'armonizzazione anche rispetto alle indicazioni europee e alle modifiche intervenute in questi anni, che hanno reso incerto e confuso l'intero piano normativo. L'armonizzazione dev'essere ispirata al principio della semplificazione, ossia alla riduzione complessiva della mole normativa. Questa riforma è nevralgica non solo per il PNRR, ma per il processo complessivo di modernizzazione del Paese e di uso delle risorse pubbliche per la crescita e lo sviluppo, per la centralità del tessuto imprenditoriale. Il Governo agisca velocemente, spero senza alcuna funzione di supplenza di altri organi,

primo luogo, si tratta di un intervento che si è reso necessario per adeguare la normativa interna al diritto europeo ed evitare così le procedure di infrazione. Si badi bene: è un adeguamento che non è una mera questione astratta, ma ha importanti conseguenze pratiche. Sono molti, infatti, i problemi applicativi sorti a seguito dell'approvazione del codice degli appalti del 2016 e delle relative disposizioni integrative e correttive dei vari provvedimenti legislativi che nel tempo, anche se ispirati dall'esigenza di assicurare la coerenza dell'ordinamento nazionale con quello comunitario, hanno in parte derogato - in alcuni casi, anche in maniera permanente - alla disciplina contenuta nel codice dei contratti pubblici. La perdita progressiva dell'omogeneità dell'iniziale intervento del 2016 non ha fatto che acuirsi con l'emergenza epidemiologica e con i successivi interventi normativi, spesso d'urgenza, che si sono susseguiti nel corso di questi ultimi due anni. Dunque, lo scopo della legge delega che ci apprestiamo a votare ha questa *ratio* complessiva: restituire alle disposizioni codicistiche semplicità e chiarezza di linguaggio, riducendo e razionalizzando le norme sul punto. La seconda ragione dell'adozione di questa riforma rientra a pieno titolo tra gli impegni recentemente assunti dal Governo con il PNRR e che necessitano di interventi celeri e contingenti nel tempo. Presidente, tre sono le linee direttrici seguite dalla legge delega in materia di contratti pubblici: intanto, norme più semplici e chiare per assicurare efficienza e tempestività nell'affidamento, nella gestione e nell'esecuzione di contratti e concessioni; luogo, tempi certi per le procedure di gara per la stipulazione dei contratti e la realizzazione degli appalti, comprese le opere pubbliche, che dovranno essere che dovranno essere sempre più orientate all'innovazione e alla sostenibilità; infine, rafforzamento della qualificazione e specializzazione del personale operante nelle stazioni appaltanti. Si tratta di obiettivi ambiziosi, ma imprescindibili per l'efficiente realizzazione delle infrastrutture e il rilancio dell'attività imprenditoriale del nostro Paese, e irrinunciabili, se si vuole concretamente garantire la piena ripresa dell'economia italiana dopo la pandemia da Covid-19. In Commissione lavori pubblici abbiamo cercato di concentrare il nostro lavoro su poche, ma mirate modifiche. Voglio precisare che si tratta di interventi che hanno trovato una sinergia condivisa fra le diverse forze di maggioranza, a testimonianza del fatto che il lavoro parlamentare può e dev'essere un arricchimento migliorativo. Ringrazio per questo i relatori, il senatore Cioffi e la senatrice Pergreffi, nonché la vice ministra Bellanova ed il ministro D'Incà per la disponibilità al dialogo dimostrata durante tutto il corso dei lavori, ma anche per le integrazioni e le modifiche concesse. Tra le modifiche più rilevanti, voglio ricordare l'attenzione mostrata al tema della sostenibilità ambientale. Abbiamo approvato misure volte a garantire il rispetto dei criteri di responsabilità energetica e ambientale nell'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, attraverso la definizione di criteri ambientali minimi da rispettare obbligatoriamente e differenziati per tipologia di importi di appalto. In merito al tema della sostenibilità sociale, invece, abbiamo predisposto misure che favoriscono la partecipazione delle piccole e medie imprese alle procedure d'appalto. Ricordo, in particolare, la previsione della possibilità di procedere alla suddivisione degli appalti in lotti e del divieto di accorpamento artificioso. Di enorme importanza, sempre grazie al lavoro emendativo, è la norma che impone alle stazioni appaltanti l'obbligo di inserire nei bandi di gara un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta. Si tratta di una modifica significativa e indispensabile. La pandemia ci ha dimostrato come il quadro economico e sociale di un Paese possa mutare rapidamente da un momento all'altro. Significa prestare attenzione all'equilibrio contrattuale, soprattutto in un settore cruciale come quello dei contratti pubblici. Il lavoro in Commissione è andato anche in un'altra direzione, quella dell'attenzione verso il lavoro e la tutela dei lavoratori. Abbiamo predisposto misure che escludono la possibilità di effettuare - in sede di offerta - ribassi relativamente ai costi della manodopera e della sicurezza, prevedendo l'applicazione delle medesime tutele economiche e normative per tutti i lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, siano essi in subappalto o dipendenti dell'appaltatore. Nello stesso solco si muove anche la misura che prevede - mediante l'inserimento nei bandi di gara - specifiche clausole volte a garantire la stabilità occupazionale e a promuovere con meccanismi e strumenti di premialità le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa. Importante è anche l'emendamento alla legge delega che impone, negli appalti di servizi sociali e della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, come criterio di aggiudicazione, solo quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa e quello che semplifica le procedure di pagamento da parte delle stazioni appaltanti, riducendo gli oneri amministrativi a carico delle imprese. Concludo, Presidente, con un accenno ai soggetti che saranno coinvolti nell'adozione dei decreti legislativi. Sugli schemi di decreti legislativi elaborati dal Governo sarà acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Ove il parere di queste ultime non sia favorevole, il Governo potrà trasmettere nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e le sue motivazioni e le Commissioni parlamentari potranno esprimere il loro parere entro un tempo di dieci giorni. Resta ferma invece, in via facoltativa, la competenza del Consiglio di Stato sulla stesura dell'articolato normativo, anche avvalendosi di magistrati del TAR, esperti esterni e avvocati dello Stato

anzi, oggi ancor di più, trattandosi di un'attività normativa che richiede competenze specialistiche altamente qualificate, appunto, come quelle dei magistrati del Consiglio di Stato. Per tutti questi motivi,

onorevoli colleghi, quella che ci apprestiamo a votare è una riforma che Fratelli d'Italia ha nelle proprie corde da tempo. La necessità di rivedere la normativa in materia di appalti era infatti diventata improcrastinabile e negli anni la stratificazione della disciplina ha generato caos interpretativo, oltre a costituire un freno allo sviluppo infrastrutturale e, in sostanza, un ostacolo alla piena realizzazione della concorrenza tra piccole e medie imprese. Avevamo dunque accolto con favore l'iniziativa di questa legge delega, riponendo su di essa speranze tangibili; una delega che peraltro risponde e si iscrive nella logica della semplificazione, così come declinata nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Sarebbe dunque stata una buona occasione per mettere alla prova la nostra capacità di sintesi e di mettere a sistema le esigenze di tutti gli attori che operano nel settore degli appalti pubblici. Fratelli d'Italia l'aveva interpretata con questo spirito in Commissione, ritenendo fondamentale accogliere le suggestioni del mondo del pubblico, e voglio ringraziare per questo gli enti locali che, per il tramite delle associazioni di categoria, hanno saputo dare in audizione un grande contributo. Contestualmente, abbiamo inteso dare spazio - nelle nostre rielaborazioni - all'altrettanto fondamentale bagaglio esperienziale del settore privato, dell'ANAC, del mondo accademico e della magistratura, perché le diverse sensibilità che ai vari livelli operano nel quadro dell'evidenza pubblica avrebbero dovuto portare un contributo essenziale, proprio nell'ottica della semplificazione. Ebbene, il lavoro fatto da Fratelli d'Italia nella gestione dell'attività emendativa a questo disegno di legge è andato esattamente in questa direzione: abbiamo analizzato i contributi di tutti, traendone le dovute conseguenze e formulando le più opportune riflessioni. Tuttavia, le grandi aspettative di cui ci eravamo caricati sono rimaste deluse da un atteggiamento della maggioranza e soprattutto del Governo, che ha sostanzialmente tradito il senso stesso della delega, determinando un'occasione persa.

Con la nostra attività emendativa abbiamo tentato di mettere dei paletti al potere legislativo delegato, sia con riferimento a determinati principi che, ad esempio, abbiamo tentato di specificare, sia con riferimento alla modifica di taluni istituti. Abbiamo provveduto all'individuazione più compiuta delle esigenze di deburocratizzazione, già inserite nel disegno di legge, cercando di introdurre parametri di riferimento inserendo ad esempio esplicitamente il rimando a principi ispiratori dei decreti emergenziali del 2020 e del 2021, che stanno producendo buoni frutti in termini di semplificazione.

di evidenza pubblica e che fossero garantite correttezza, trasparenza e legalità laddove appare necessario un contestuale alleggerimento delle procedure.

avrebbe garantito che le imprese che vantano crediti certificati con le pubbliche amministrazioni non potessero essere escluse in caso di irregolarità fiscali non definitivamente accertate. contributi di buon senso, che vanno nella direzione che tutti si aspettavano. Anche quest'ultima evidenza, che è una battaglia di civiltà che impedirebbe allo Stato di comportarsi da tiranno nel momento di esigere i crediti e di essere indulgente invece con se stesso nel momento di pagare, è stata da questa maggioranza nei fatti rigettata. rigettata. Non è una questione di poco conto, né un cavillo per tecnici, perché, quando le pubbliche amministrazioni non pagano alla scadenza, le prime imprese che vanno in sofferenza sono quelle che costituiscono il nerbo dell'economia italiana, le piccole e medie imprese, che non hanno sufficiente disponibilità finanziaria e rischiano di avere, a causa delle inadempienze delle stazioni appaltanti, gli accertamenti fiscali che le escludono poi dalle successive gare, come un furioso cane che si morde la coda: oltre al danno, anche la beffa. In materia di appalti pubblici, laddove sono pregiudicate le piccole e medie imprese, è lì che dilagano non solo e non tanto le grandi concentrazioni economiche, ma anche la grande criminalità organizzata. Con questa delega così ampia, signori, non si comprende la direzione che il Governo vuole prendere per il futuro per la definizione della disciplina in materia di appalti, che possiamo solo desumere dalla natura degli emendamenti che abbiamo presentato e che ci avete bocciato. bocciato. Non è la direzione che ci piace, né quella che serve all'impresa italiana e di cui hanno bisogno le pubbliche amministrazioni per vedersi facilitato il lavoro. In conclusione, a Fratelli d'Italia premeva la revisione della disciplina in maniera organica, indirizzando il legislatore delegato e astringendolo a principi definiti, affinché fosse dato ossigeno alle imprese, strumenti agili alla committenza e garanzia di trasparenza e correttezza per la realizzazione di principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione. A noi, colleghi, non pare che questo sia avvenuto e, per quanto confidiamo che i nostri intendimenti possano essere oggetto di dibattito alla Camera e possano trovare albergo nella stesura definitiva del provvedimento, oggi esprimeremo un voto contrario: lo dico perché il clima che ho respirato e abbiamo vissuto con i colleghi della Commissione è stato davvero di totale armonia e li voglio ringraziare, a partire dai relatori. Abbiamo davvero lavorato insieme e li ringrazio per gli attestati di stima che abbiamo ricevuto anche in questa sede, che sono puntualmente ricambiati. però - e lo dico a nome di tutto il Gruppo Fratelli d'Italia - che si stia perdendo una grande occasione.

ha detto il vice ministro Bellanova, che ovviamente ringrazio per il lavoro che insieme abbiamo fatto, rispetto alla delega iniziale. Mi pare un buon esempio, di questi tempi, di come valorizzare le parole importanti che il presidente Mattarella ha detto a proposito del rapporto tra Governo e Parlamento. Di questo buon lavoro è assolutamente doveroso ringraziare i colleghi relatori Cioffi e Pergreffi

un'altra premessa, che mi sta molto a cuore per il ruolo che abbiamo svolto nella precedente legislatura, nella quale abbiamo approvato una riforma degli appalti, seguita, in particolar modo, dal ministro Delrio, che abbiamo votato e condiviso. Personalmente, su alcuni aspetti non ero del tutto d'accordo, la dialettica che si è sviluppata tra coloro i quali ritenevano quella legge perfetta e immodificabile e coloro i quali la ritenevano, invece, quasi l'origine di tutti i mali è stata sbagliata: si trattava di una buona legge, che ha dato effetti positivi, ma naturalmente i rimaneggiamenti che ci sono stati nel corso degli anni successivi hanno reso importante e inevitabile mettere mano a una riforma più complessiva, che desse nuovamente vita a un disegno unitario e non frammentato. Per questo stiamo lavorando.

norma ha a che fare con il PNRR per un altro motivo, ossia perché l'Unione europea ci ha chiesto una serie di riforme di tipo strutturale e non contingente, che ci siamo impegnati a sviluppare e ad approvare in modo tale da essere in regola con gli impegni: la riforma degli appalti, quella del fisco e quella della giustizia. Grazie al lavoro che abbiamo fatto, saremo in grado di rispettare i tempi. Già il collega Astorre, in un bell'intervento, ha segnalato una serie di emendamenti del PD che sono stati recepiti, approvati e che hanno migliorato di legge. Abbiamo fatto un ottimo gioco di squadra, a partire ovviamente dalla presidente Malpezzi e dal collega D'Arienzo. Se dovessi sintetizzare con un'unica espressione il lavoro che abbiamo fatto, direi: semplificazione, direi: semplificazione, efficienza e rapidità, ma nell'assoluto rispetto di trasparenza, sicurezza sul lavoro, diritti dei lavoratori e sostenibilità ambientale (un emendamento del collega Mirabelli in tal senso è stato assolutamente pregevole); insomma, direi la traduzione in pratica di un approccio autenticamente riformista o, almeno, di quello che noi del PD riteniamo essere il riformismo. Un emendamento particolarmente significativo, frutto del concerto tra Governo e Parlamento, è quello in materia di revisione dei prezzi, che dovrà obbligatoriamente essere sempre presente in bandi, avvisi e inviti, per essere utilizzato in particolari condizioni di natura oggettiva. Si pensi a quel che sta accadendo oggi

Certo non entrerà in vigore oggi, ma quando saranno stati approvati definitivamente la legge e i decreti attuativi; si tratta però di un segnale importante che diamo alle imprese, dicendo che ci stiamo pensando e a regime ci arriveremo.

Abbiamo lavorato su questo versante, ma non abbiamo mai dimenticato le altre questioni per noi importantissime: la trasparenza e le misure a tutela dei lavoratori e quelle relative alla sostenibilità ambientale. Non potranno essere mai fatte gare al massimo ribasso, né essere effettuati ribassi sul costo della manodopera e sulla sicurezza dei lavoratori. Le gare in materia di servizi sociali e della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica e, in genere, quelle di servizio ad alta intensità di manodopera non potranno mai essere assegnate con l'unico criterio del prezzo. Non possiamo pensare che nelle mense ospedaliere o in quelle scolastiche

fluida, scivolosa, difficile da irreggimentare e che, visto che siamo in tema di anniversari, qualche volta a me fa venire in mente una bellissima canzone di Lucio Dalla, che a un certo punto dice che il pensiero è come l'oceano: non lo puoi bloccare, non lo puoi Anche la materia dei lavori pubblici ha tante di quelle innovazioni che riuscire a comprimerla è complicato, devo dire con grande fortuna dei bravissimi avvocati che se ne occupano durante tutti i contenziosi. l'ardire e l'ambizione di irreggimentarla; abbiamo pensato, invece, di poterla valorizzare, ordinare e implementare in massima misura a vantaggio del Paese. Siamo contenti di poter dire che il Parlamento in tale direzione ha fatto la sua parte.

e stabilire i principi, è stato molto importante ed efficace. In questo mi associo anche io ai ringraziamenti a tutti i membri della Commissione, ai relatori e alla Vice Ministra,

soprattutto in un tema come quello degli appalti pubblici. Il senatore Margiotta sa che siamo intervenuti in questa materia svariate volte,

sono fiduciosa - un lavoro organico. Tutti gli interventi, che spesso sono stati non sistematici, ma asistematici, hanno prodotto una selva e una stratificazione di

ed è ancor più importante perché riuscirà a risolvere alcuni problemi applicativi che si sono riscontrati a causa della stratificazione delle norme in questo settore. Penso che si possa finalmente dare ordine a un quadro giuridico del settore che attualmente è assolutamente poco organico e chiaro.

Noi abbiamo un problema di qualificazione, in generale, della pubblica amministrazione e anche di capacità progettuale, di chiarezza dei progetti e di indicazione. Nel disegno di legge di delega sono stati stabiliti dei principi - a mio avviso -assolutamente fondamentali, come l'assoluta inderogabilità delle misure a tutela del lavoro, della sicurezza del contrasto al lavoro irregolare, quindi a tutela della legalità e della trasparenza. Una ripresa economica sana - a mio avviso - può avvenire solo e unicamente se è ben chiaro il quadro di legalità e di trasparenza in cui

a garantire il rispetto dei cosiddetti CAM, cioè i criteri ambientali minimi, che sono un elemento non di

previsti la facoltà e l'obbligo, tra l'altro, per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti tutte le specifiche clausole sociali. Inoltre, l'utilizzo del massimo ribasso è assolutamente escluso se non con delle tipizzazioni molto precise, con l'esclusione di alcuni settori. Ha fatto bene il collega Margiotta a dare

sono stati rispettati. Noi contiamo - e lo dico al Governo - non solo di vedere presto i decreti legislativi, perché è assolutamente importante che siano subito portati all'attenzione del Parlamento, ma anche che questa volta, proprio in omaggio e in coerenza con il buon lavoro che è stato svolto

vorrei ringraziare i colleghi della Commissione e il vice ministro Bellanova, con la quale abbiamo lavorato in queste settimane per licenziare un provvedimento importante. È una legge delega torneremo ad esprimere dei pareri, ovviamente, ma l'indirizzo del Parlamento è fondamentale ed è quello su cui abbiamo voluto fissare la nostra attenzione. Prima ci siamo dati, delle regole. Le regole sono il Parlamento dà degli indirizzi, che poi dibatte al proprio interno, all'interno della Commissione, che rappresenta, quindi, tutti i Gruppi parlamentari. Il primo obiettivo era quello di capire se c'era la volontà, se c'era l'intento di trovare una sintesi, una soluzione che andasse nell'interesse generale.

il pensiero di fissare degli obiettivi che scaturivano da necessità oggettive. C'era il problema della rapidità degli appalti;

forse sarà meglio non eseguirli. Come qualcuno ha detto, se abbiamo già fatto degli accordi quadro, magari due anni fa, vuol dire che, anziché fare 200 chilometri di asfalto, ne realizzeremo 80.

essere conseguente all'aumento dei prezzi, ma non possiamo infinitamente seguire questo filone. filone. Una volta fissato il concetto che il Parlamento aveva il diritto e la necessità di esprimere un punto di vista e di dare indirizzi chiari al Governo, abbiamo parlato col Governo, che ha accolto questo punto di vista.

meno. Il vice ministro Bellanova, che è politica di lungo corso, queste cose le capisce al volo. Magari, la tecnicità di qualche Dicastero

ringraziare l'intuizione del relatore Cioffi. Io definivo l'argomento come la necessità di coinvolgere le imprese del territorio nei lavori che si sviluppano sul territorio. L'uomo, più acculturato e di mestiere, ci ha suggerito la definizione di *small business act*, che è conseguentemente il concetto della direttiva europea che tiene conto della territorialità delle piccole e medie imprese.

per scegliere l'impresa, perché così era previsto in una delibera della Giunta regionale pugliese. Ebbene, questo concetto ormai l'abbiamo superato, perché abbiamo tolto di mezzo il sorteggio nella scelta delle imprese. Guardate che è un fatto epocale

quindi la nazionalità di quello che facciamo: le piccole imprese, il territorio, la revisione dei prezzi, i nostri Le coperture assicurative per i professionisti sono un altro elemento importante: se fai l'ingegnere, il geometra o l'architetto, come allunghi la penna subito qualcuno ti dà una botta sulla mano, perché pagherai personalmente per te, i figli, i nipoti, i cugini e gli zii. coperture è un fatto veramente importante. Le fideiussioni a scalare sono una cosa incredibile. Se uno faceva un appalto da 10 milioni, rimaneva impegnato, nonostante gli stati di avanzamento, per 10 milioni fino alla fine dell'opera: una follia significava impedire all'impresa di andare avanti su altri lavori, perché magari il castelletto che aveva l'impresa non era sufficiente per coprire l'impegno fideiussorio. Si tratta quindi di un altro elemento epocale che le imprese aspettavano.

Siamo tutti d'accordo che non siamo d'accordo Vice Ministro, sta quindi a lei il compito di trasmettere il fatto che siamo d'accordo perché non siamo d'accordo.

a condizionare le scelte sui lavori pubblici, sugli appalti e sulla vita istituzionale di questo Paese.

Noi siamo a disposizione per trovare un accomodamento, in ogni caso. Forza Italia vota convintamente il provvedimento in esame perché rispecchia un punto di vista che portiamo avanti da vent'anni e che con questa approvazione probabilmente va nella direzione giusta. Quindi, grazie a tutti e buon lavoro.

tutta l'8a Commissione che si è impegnata in questo provvedimento abbastanza particolare e adesso spiegherò anche il perché. Quella del codice dei contratti è una storia tutta da scrivere ed è una storia infinita. Il codice dei contratti, quello di cui stiamo parlando e di cui parliamo quasi quotidianamente, è riferibile al decreto legislativo del 18 aprile 2016, Il codice si era reso necessario perché era uno strumento che doveva recepire le direttive europee nn. 23, 24 e 25 del 2014. l'obiettivo finale era quello di garantire valori fondamentali come la flessibilità, la trasparenza, la prevenzione della corruzione, delle infiltrazioni della criminalità organizzata, introducendo - rispetto alle direttive europee - ulteriori strumenti e anche istituti inediti improntati a un maggior rigore, senza però cadere nel *gold plating*, la pratica di introdurre livelli di regolazioni superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive.

Questo cambio di approccio aveva lo scopo di garantire una maggiore semplicità e una maggiore snellezza.

invece di adattarsi alle direttive europee, il Parlamento riuscì, con una legge del 28 gennaio 2016, la n. 11, recante deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive nn. 23, 24 e 25

venne sostituito con quello del 2016, che doveva recepire queste direttive. Dal 2014, queste direttive non sono ancora state recepite, nonostante ci sia stata un'attività legislativa tesa alla semplificazione e al riallineamento di queste procedure che non è mai avvenuta. Siamo nel 2022

una visione del codice come di un compendio normativo finalizzato esclusivamente ad alleggerire, semplificare e rendere chiare

tutta la normativa riferibile al tema - riportandoci alla normativa europea rispetto alla quale altri Paesi sono molto più avanti di noi dal 2014 proponendo, magari, uno strumento che, oltre a recepire, poteva fare un passo in più e arrivare alla condizione di rivedere quello che è il compendio normativo stesso, in modo tale da offrire agli operatori e a coloro che fanno uso quotidianamente di questo codice uno strumento veramente efficace e soprattutto immediato.

declinare principi e regole che si trascinano da molti anni. Sono regole che avrebbero dovuto trovare la loro attuazione già precedentemente. Se oggi chiediamo a qualcuno come usa il codice, sa che una parte è stata sospesa per l'intervento del provvedimento sblocca cantieri (solo fino al sotto soglia); si è andati in deroga ed è intervenuta un'altra cosa; per cui a spizzichi e bocconi si è smantellato anche l'impianto di questa normativa al punto tale che si è creata una condizione di confusione impressionante.

non verranno emanati i decreti attuativi, questo regolamento, con tutto lo sforzo e il lavoro che è stato fatto dalle Commissioni, resterà qui.

che è quasi dentro casa, e non più alle porte; una situazione sociale difficilissima; un concetto di pace che si sta allontanando. Se vogliamo essere operativi e veramente

succeda di nuovo. Nel 2022 siamo ancora qui a riallinearci a vecchie situazioni che non sono state prese in considerazione: è l'ultima *chance* che abbiamo. Dopodiché, le nostre imprese, i nostri operatori, tutti i soggetti interessati da queste misure si troveranno nelle condizioni di non poter essere operativi. E non essere operativi, in costanza di situazioni così drammatiche, significa non dare la possibilità all'Italia di riprendersi e di attuare quello per cui noi

Signor Presidente, colleghe, colleghi, componenti del Governo, Ministro - arrivato giusto in tempo per la mia dichiarazione di voto - nell'annunciare favorevolmente il parere parere del MoVimento 5 Stelle al provvedimento al nostro esame, devo dire però a tutti i miei colleghi che noi oggi siamo qui impegnati per dare un segnale concreto al Governo:

come quello sul codice dei contratti, noi in Commissione siamo stati capaci di trovare una convergenza molto larga e trasversale. Ciò sta a significare che, quando al centro del dibattito ci sono gli interessi dei cittadini, è possibile tranquillamente andare oltre le problematiche che esistono tra di noi, pur partendo da visioni originate in contesti molto diversi, come diceva prima il senatore Mallegni. Si privilegia l'offerta economicamente più vantaggiosa, quando invece noi vorremmo privilegiare altro, contestualizzando la modalità di aggiudicazione.

fa. Bastasse solo quello. Dobbiamo anche recepire la normativa europea e, quindi, la complessità aumenta talmente tanto che gli operatori del settore hanno estrema difficoltà a rincorrere le modifiche del codice degli appalti. E questo ci sembra molto chiaro. E questo ci sembra molto chiaro. È però anche vero che l'Italia, a differenza di altri Paesi, ha un riconoscimento storico nella qualità delle sue maestranze edili. In Italia noi facciamo impresa di costruzione.

all'ultima legge quadro, il decreto legislativo n. 50 del 2016, i cui regolamenti attuativi si sono persi nel nulla. È questo il problema del fallimento di quel codice. *(Applausi)*. Per tale motivo noi abbiamo dovuto incidere sulla materia durante il corso di questa legislatura, cari colleghi, a iniziare con il decreto-legge Genova. sblocca cantieri abbiamo fatto qualcosa di formidabile. Oggi cambiamo l'aggettivo, lo spostiamo da più basso o, al massimo, se parliamo di prezzo oppure di ribasso. È però anche vero che vero che noi dobbiamo cercare di agevolare procedure tarate in base all'obiettivo da perseguire. Se quell'obiettivo ha una tecnologia molto convincente, allora è premiante - come diceva il senatore Mallegni - l'offerta economicamente vantaggiosa. Altrimenti - come avvenuto con lo sblocca-cantieri - finalmente il prezzo più basso ce lo siamo messi alle spalle definitivamente, nominando finalmente il prezzo più congruo. *(Applausi)*. Siamo poi arrivati alla fine a intervenire con il decreto-legge semplificazioni nel corso dell'anno 2020, praticamente ieri. Ora però è il momento di accelerare la normativa sui lavori perché stanno arrivando i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Sono fondi preziosi che ci aspettano. con i Gruppi parlamentari abbiamo posto l'accento sull'accelerazione dell'attuazione dei lavori pubblici. Attenzione: attuazione. Cerchiamo di superare il concetto della mera realizzazione. Per realizzare un intervento bisogna partire dalla pianificazione, dalla programmazione, dalla progettazione; poi ci sono la gara, l'affidamento, l'inizio dei lavori, la realizzazione, la manutenzione, il collaudo

quelle della progettazione e di affidamento dei lavori. Certo, si stima che con il PNRR siano 100 i miliardi che verranno appaltati. Adesso però il Governo deve avere il coraggio di gettare il cuore oltre l'ostacolo, perché oltre a quei lavori pubblici ci sono centinaia di miliardi di lavori edili privati. Al riguardo, in Commissione stiamo discutendo di un disegno di legge per la delega al Governo sul riordino di tutta la normativa sulle costruzioni. Vorrei ricordare a tutti che il settore dei lavori edili

distinguere nettamente la regolamentazione tra lavori pubblici, servizi e forniture, perché sono argomenti troppo diversi per essere trattati in maniera univoca. Spero che il Governo lo possa fare attraverso i regolamenti attuativi. Volevamo proteggere maggiormente i subappaltatori: sentiamo parlare di crisi di impresa ma, quando l'appaltatore principale ha una crisi o fallisce o ha dei problemi economici e non ha avuto ancora i soldi da parte dello Stato, proponevamo di far subentrare lo Stato far subentrare lo Stato a sostegno di quel fornitore o di quel subappaltatore. Allo stesso modo, volevamo agevolare la procedura di aggiudicazione con il criterio della media delle offerte, col metodo anti turbativa e con la disciplina del taglio Volevamo inoltre privilegiare, con i dignitosi compensi che sono dovuti, le consulenze esterne quando le pubbliche amministrazioni non ce la fanno a progettare.

quelle che il mondo ci invidia, attraverso una somma che poteva essere allocata all'interno del quadro economico. Non è stato così. Ma vi diciamo che non smetteremo di combattere su questi temi, perché non ci arrendiamo.

e anche per il compenso che deve essere garantito a queste persone che lavorano dalla mattina alla sera e sostengono degli sforzi enormi, certe volte lontano dalle proprie case. Abbiamo escluso dalle somme previste dal ribasso di gara gli importi relativi ai costi per la manodopera e la sicurezza. *(Applausi)*. tutela delle imprese, delle piccole e medie imprese, prevedendo la suddivisione in lotti con criteri qualitativi e quantitativi, e meno male che lo abbiamo fatto.

a carico dell'amministrazione appaltante, quindi a carico dell'ente pubblico, che copre i rischi professionali del professionista. Abbiamo garantito la centralità di questo Parlamento. Come è stato detto da tanti colleghi che mi hanno preceduto, il Governo deve ascoltarci. Noi porremmo delle condizioni, se servono. Se il Governo non le vuole accettare, ci deve venire a spiegare il perché. *(Applausi)*. Mi sembra veramente una presa di posizione importante da parte di questo Parlamento, troppe volte tartassato e superato da decreti-legge. Infine, forse uno dei punti più importanti - sicuramente lo è per me - riguarda il perseguimento della transizione ecologica. Abbiamo detto chiaro e tondo che negli appalti bisogna rendicontare l'obiettivo energetico ambientale

Grazie,

Non avevo dato alcun numero, senatrice.

Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, prendo la parola per portare in quest'autorevole Aula la voce dei pescatori pescatori della storica marineria di Marina di Schiavonea, nella mia città, Corigliano-Rossano. Porto anche la voce dei pescatori di Cariati, Crucoli, Cirò Marina e Crotone e di tutti i pescatori calabresi e italiani. Raramente i pescatori chiedono o si fermano. Loro, il popolo del mare, sono abituati alle difficoltà e alle tempeste, quindi se in questi giorni si sono fermati e manifestano è per una ragione sacrosanta. L'aumento esponenziale del carburante non consente più ai pescatori italiani di uscire in mare, come si dice in gergo, attendere e proseguire la loro attività che costituisce il primo anello fondamentale di un'importante filiera per tutta l'economia nazionale e che dà lavoro a tantissime famiglie. Gli armatori non ce la fanno più a sostenere le spese del gasolio, che è aumentato quasi del 60 per cento, e andare a pescare in questo momento accumulerebbe solo debiti e non guadagni. Tutto questo ha come conseguenza la perdita di reddito di tante e tante famiglie. E allora, presidente Draghi, ascolti le ragioni e le esigenze dei pescatori e le sostenga con strumenti che lei, grande esperto di economia e finanza, saprà ben trovare, saprà ben definire, e saprà ben aiutare, con tali strumenti, i pescatori che in questo momento invocano aiuto. Pensi ad un necessario scostamento di bilancio se è il caso, perché siamo in una situazione estrema, siamo in guerra, in un momento in cui aumenta il prezzo delle materie prime. Al ministro Patuanelli e al sottosegretario con delega alla pesca Battistoni dico di non girare più la testa come sta avvenendo in questi ultimi tempi: difendete e sostenete i pescatori nella loro legittima e seria richiesta d'aiuto. I pescatori, con la dignità e la riservatezza che li ha sempre contraddistinti, non possono e non devono essere abbandonati a se stessi. Mi auguro che presto ci saranno riscontri positivi per rivedere i nostri pescherecci solcare di nuovo il mare. *(Applausi)*.

Signor Presidente, un ennesimo femminicidio ha macchiato di rosso le pagine di cronaca di questi giorni, a Pontecagnano, in provincia di Salerno. Questa volta la vittima si chiamava Anna Borsa e aveva appena trent'anni. Stava lavorando Anna, nella parrucchieria dove era impiegata, quando il suo assassino l'ha raggiunta e le ha sparato a sangue freddo un colpo alla tempia. La giovane donna è morta immediatamente e in un attimo tutti i suoi sogni sono stati spazzati via. Ancora una volta ad uccidere è un ex fidanzato che non accetta la fine della relazione. Ancora una volta ad uccidere le donne sono uomini che hanno bisogno di imporsi con la violenza, uomini che dicono di amarle e invece le ammazzano. I casi di violenza sulle donne in Italia raggiungono ancora numeri allarmanti. Questo Parlamento ha dato, nel 2019, un importante segnale con l'approvazione del codice rosso, ma purtroppo non è abbastanza. Sono ancora troppi i casi in cui le donne non sono libere di compiere le proprie scelte senza temere per la propria vita. Non dobbiamo vergognarci nell'ammettere che in questo Paese le donne sono ancora troppo spesso relegate a ruoli subalterni e che fino a pochi decenni fa era la normalità. Dobbiamo riconoscere i limiti della nostra società per poterli superare. Gli uomini per primi devono essere al fianco delle donne perché si possa davvero sperare nel cambiamento. Dobbiamo intervenire per affrontare il problema alla radice ed educare gli uomini affinché rispettino le donne. Ognuno di noi deve farsi carico del dolore che la violenza genera, perché il male che affrontiamo è un male sociale, un male profondo che affonda le sue radici nella nostra cultura ancora troppo maschilista. Lo dobbiamo alle vittime incolpevoli, alle loro famiglie, alle comunità sconvolte dalla brutalità di questi gesti a cui oggi rivolgo tutta la mia commozione e il mio cordoglio.

Presidente, onorevoli colleghi, nella condanna unanime della sanguinosa guerra in Ucraina, scatenata dall'aggressione delle forze sovietiche, voglio ringraziare l'intera collettività del nostro Paese, che ancora una volta sta dimostrando il suo profondo spirito di solidarietà ed il suo forte senso umanitario *Open Arms*: a braccia aperte. Esso rappresenta, in questa come in tantissime altre occasioni, la dimostrazione evidente che il popolo italiano ha uno spirito comunitario e solidale verso chi è in difficoltà e ha bisogno di aiuti concreti, di una mano tesa, al di là delle diverse posizioni o dei differenti modi di interpretare la crisi in Ucraina. La guerra di aggressione non ha colore politico o convinzione religiosa. Va sempre, ovunque e comunque condannata, senza se e senza ma. Rappresenta la negazione della stessa natura umana. A braccia aperte, con l'animo gonfio di dolore, si sono moltiplicate le iniziative spontanee di associazioni solidali, di singoli cittadini, di intere famiglie, di attività commerciali, con l'invio di prodotti alimentari, farmaci, mezzi di prima necessità, coperte, vestiario per aiutare la popolazione civile, bambini, donne e anziani, vittime innocenti di una guerra che non volevano, ma di cui pagano le conseguenze più drammatiche. Lo spirito comunitario e il rispetto della vita umana certamente non si possono fermare solo a tutto ciò. Solidarietà senza frontiere: ecco il profondo spirito solidale, l'accoglienza dei profughi nelle nostre città, nelle nostre parrocchie, nelle nostre comunità. Esseri umani indifesi che, stremati dalla stanchezza, dai digiuni, dalle sofferenze fisiche, con i cuori affranti dal distacco dei loro affetti, dai loro cari e dagli orrori della guerra, che li ha costretti a fuggire dalla loro terra natia, sono già nel nostro Paese; e tanti altri ne stanno arrivando, come d'altronde negli altri Paesi europei. Si calcola che, allo stato, sono circa due milioni i profughi già fuggiti dall'Ucraina che brucia. Gli orrori della guerra, il dolore di chi soffre, le violenze sui loro corpi, gli sguardi impauriti rappresentano un dramma epocale per tutti noi. Questa tregua occorre affrontarla tutti insieme, con profondo spirito di solidarietà, che va oltre il singolo cittadino, ma anche oltre la singola comunità o il singolo Paese. Dobbiamo tendere una mano a chi chiede aiuto. Questo è lo spirito, profondamente cristiano, umanitario e anche veramente europeista. Il nostro animo triste e addolorato deve reagire e aprirsi, superando confini geografici e barriere culturali. Apriamo i corridoi umanitari veri, per salvare vittime innocenti. La voce del dialogo sia più forte del crepitio delle mitraglie e dello scoppio delle bombe. Non più carnefici e vittime, ma una tregua immediata per avviare un dialogo vero di pace. *(Applausi)*.